L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

si è costituito qualche settimana fa e abbiamo anche saputo dal presidente Fini che dopo il voto di fiducia questo Gruppo parlamentare sarebbe passato all'opposizione.

le dichiarazioni - debbo dire - irricevibili del senatore Gasparri a proposito della tecnica che le forze di polizia dovrebbero usare

ripeto con parole mie, ma il senso era molto chiaro - l'arresto preventivo di quegli studenti che si suppone possano intervenire in modo non pacifico nella prossima manifestazione. Signor Presidente, a parte ricordare che non c'è un solo costituzionalista, tra quanti si sono espressi sull'argomento, che non abbia rilevato l'assoluta incostituzionalità della proposta, a parte rilevare che anche le stesse rappresentanze delle forze di polizia hanno preso vistosamente le distanze dalla proposta del senatore Gasparri, vorrei vorrei ricordare all'Assemblea che i senatori del Partito Democratico avevano chiesto che questi nostri lavori sulla riforma universitaria venissero rinviati

signor Presidente, che gettare benzina sul fuoco non sia un atteggiamento responsabile. Penso che dobbiamo che dobbiamo colloquiare con la protesta studentesca, dobbiamo condannare in modo chiaro ed esplicito ogni violenza, ma dobbiamo sapere che nella protesta ci sono molte questioni che il Parlamento ha il dovere di esaminare e ci sono molte risposte che il Parlamento ha il dovere di dare ai ragazzi che scendono in piazza per protestare contro la riforma universitaria. Ritengo sia un azzardo un azzardo grave e una provocazione grave che addirittura da parte del Capogruppo del partito di maggioranza venga richiamata la necessità, da parte della polizia, di arrestare gli studenti che non sono d'accordo con la riforma e che scendono in piazza, violando in questo modo tutti i diritti dei cittadini che sono tutelati dalla nostra Costituzione. Signor Presidente, la prego di riferire anche al presidente Schifani le mie osservazioni, e la ringrazio per avermi concesso la parola.

Presidente, colleghi, anch'io, a nome del Gruppo Italia dei Valori, ho la necessità di intervenire

si va surriscaldando, certamente non per colpa degli studenti che protestano. La protesta è legittima...

al riguardo l'opinione è condivisa dall'Italia dei Valori - che questa riforma ruba il futuro alla ricerca, all'università, ai giovani e al Paese! Questa è la realtà. PdL)*. Dire che ci sono tra gli studenti dei potenziali assassini altro non significa che voler far sorgere un incidente grave perché il Governo, che è debole, deve necessariamente avere

infatti, da una maggioranza raccogliticcia e d'accatto ed evidentemente il Paese ha capito in che direzione vuole andare.

vorrei infatti che in questo modo si perpetrasse un vizio del nostro costume politico, quello cioè di mettere sul banco degli accusati

noi siamo per il confronto fino in fondo sulle motivazioni che sono alla base del provvedimento.

quindi nessuna volontà di criminalizzare le argomentazioni e le critiche alla riforma. Crediamo, però, di dover affermare attraverso questo atteggiamento tre semplici questioni, che derivano anche dalla storia di questo Paese, e in particolare dalla storia dei movimenti studenteschi, che conosco bene.

tutelata sempre e comunque: lo chiediamo a chi entra in questo Paese come ospite, dobbiamo chiederlo innanzitutto a chi è cittadino di questo Paese. *(Applausi dal di per sé, una scriminante. Se si afferma questo, si è cattivi maestri. In passato è già avvenuto, ed è un errore che non dobbiamo ripetere. In secondo luogo, la responsabilità è personale, in capo ad ogni singola persona e ad ogni singolo individuo. Nessuno pensa di criminalizzare movimenti, ma laddove ci sono atti contrari alla legge, come ci sono stati nei giorni passati, questi atti devono essere denunziati per quello che sono; partecipare ad un movimento non vuol dire poter fare quello che si vuole e addebitarlo poi al movimento. In questo modo, si finisce infatti per scaricare sul movimento le proprie responsabilità; richiamare la responsabilità personale è anche un modo per difendere i tanti ragazzi che in buona fede sono contro la nostra riforma.

È uno dei modi per poter gestire situazioni come queste. Come i colleghi della sinistra sanno, prevenire anziché reprimere è un vecchio *refrain* che si è sviluppato proprio nell'ambito della sinistra, sin dai tempi della sinistra storica; sono nati e caduti Governi della sinistra storica su questa base. L'attività di prevenzione, collega Zanda, è prevista dal testo unico di pubblica sicurezza: nessuno chiede che si vada oltre quello che è previsto dalle attuali leggi e dall'attuale testo unico.

che il Parlamento possa cedere di fronte alle azioni non commendevoli che abbiamo visto nell'ultima manifestazione, perché far questo vorrebbe dire venir meno alla nostra funzione ed incoraggiare quelle frange violente che hanno già avuto modo di esprimersi. Noi questa responsabilità non ce la prenderemo. Saremo responsabili fino in fondo ed è anche per questo che vogliamo approvare ora e in tempi rapidi, dopo un'ampia discussione, questa riforma. I colleghi dell'opposizione sanno, perché l'hanno vista nascere all'interno della Commissione, che questa riforma non merita di diventare il simbolo e il simulacro di una crisi più profonda. Nessuno ignora che la crisi più profonda c'è, ma quando i provvedimenti parlamentari si caricano di un significato improprio, non si fa un buon servizio né al Parlamento né ai giovani che contro quei provvedimenti si scagliano. Riportiamo la

Signor Presidente, noi siamo convinti che il diritto a manifestare deve essere sempre garantito a tutti: al riguardo non vi sono dubbi. Siamo anche convinti, però, che contro i violenti

dal magistrato buonista di turno. Ha fatto bene, dunque, il ministro Alfano ad inviare gli ispettori. Per quanto riguarda la prevenzione, siamo convinti che sia giusto intervenire da questo punto di vista.

la discussione che si avvia oggi sulla riforma e il dibattito che si è aperto qualche giorno fa con l'informativa del ministro Maroni sul tema della sicurezza delle manifestazioni e sul modo in cui le le forze dell'ordine devono concorrere a garantire che il principio costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero possa essere garantito

medesimo invito anche ai parlamentari che parlano fuori quest'Aula. Infatti, ho ascoltato dichiarazioni irresponsabili, che possono riguardare un dibattito che avrà la sua sede parlamentare propria, cioè le Commissioni

deve esercitata da tutti: in quest'Aula a cominciare dai colleghi dell'Italia dei Valori, fuori da quest'Aula da altri colleghi della maggioranza, che farebbero bene ad abbassare i toni e a non incrementare, con dichiarazioni avventate,

Presidente, ho un quesito da rivolgere alla maggioranza e al Governo. Si vuole approvare in quest'Aula la riforma dell'università? Si vuole ricercare il consenso dei senatori ed eventualmente registrarne i dissensi nel merito? si vuole fare di questo dibattito parlamentare l'occasione per uno scontro politico ricercato a tavolino? Questo è il tema. il tema. Abbiamo iniziato la fase politico‑parlamentare nella quale ci troviamo con un discorso svolto in quest'Aula dal Presidente del Consiglio, il quale si è rivolto, per ottenere la fiducia, ai moderati e alla moderazione.

colleghe e colleghi senatori, in occasione dell'intervento del Ministro dell'interno, quel giorno ci siamo pronunciati tutti, sono chiare le posizioni di tutti,

Voi, colleghi della maggioranza, ci volete portare a un dibattito sull'università, o immaginate di travolgere il merito della odierna discussione per rispondere alla piazza e alla sua componente estremista, anziché riportare qui

Allora, se in quest'Aula, a nome del Gruppo del PDL, si fa, cari colleghi, un intervento di richiamo alla responsabilità, siamo pronti a condividerlo.

Non ho simpatia per i magistrati politicamente schierati, ma proprio per questo non li identifico come tali quando esercitano il loro lavoro. La mia conclusione è questa. Siccome in Aula ci si richiama spesso alla serenità, alla legalità, al dovere di tutti di essere in condizioni di promuoverle al di fuori di quest'Aula e di non fare qualcosa che determini conseguenze negative al di fuori vorrei pregare chi ha parlato a nome del Gruppo del PdL fuori di qui di rivolgersi ai commercianti della Capitale, agli operatori economici, alle famiglie, e di chieder loro se per caso la minaccia di assassinii... ...per le strade sia bene accetta a coloro che si aspettano, dopo un anno di grandi difficoltà economiche, che la piazza sia tenuta responsabilmente in equilibrio, sotto il controllo delle forze dell'ordine, e non venga incendiata da coloro che irresponsabilmente vogliono continuare a dichiararsi moderati e poi ad essere degli estremisti. Questo è un tipo di responsabilità che, mi auguro, colleghi della maggioranza, dopo questo dibattito preliminare suscitato dal collega Zanda si interrompa qui e nelle dichiarazioni che fate fuori dal Parlamento, perché non potete venire a farci la predica prenatalizia, come ha fatto il collega Quagliariello, e, appena uscite davanti alle telecamere,

disegno di legge e non ha potuto raggiungere le condizioni per esprimere un mandato al relatore, senatore Valditara.

Noi abbiamo chiesto di poter lavorare nella settimana precedente il voto del 6 e del 7 dicembre sulla legge di stabilità, ma non vi è stata la possibilità di operare in Commissione perché non si è raggiunta l'unanimità, essendo quei giorni ancora vincolati, come da Regolamento, dalla sessione di bilancio.

a luglio dal Senato non era stato in nessun modo cambiato e che la Camera aveva quindi operato essenzialmente integrando con alcuni

Commissione, cioè nel pomeriggio, abbiamo stabilito il calendario dell'impegno in Commissione ed avremmo dovuto terminare

Gli emendamenti presentati entro le ore 20 del giorno 15 erano stati 538, ed al riguardo devo ringraziare davvero gli Uffici della 7a Commissione per il lavoro di riorganizzazione di questi emendamenti, che ha richiesto buona parte della nottata tra il 15 e il 16.

da esaminare e votare altri 503: un numero esorbitante rispetto alle ore a disposizione. Si è chiesto alle opposizioni se non ritenessero di poter ritirare gli emendamenti, onde procedere al al voto del mandato al relatore. Le opposizioni si sono dichiarate favorevoli al ritiro degli emendamenti, purché tre o quattro emendamenti venissero

però la disponibilità a ritirare tutti gli emendamenti, tenendo conto che la Camera aveva introdotto 55 modifiche e noi chiedevamo tre modifiche sostanziali, che probabilmente avrebbero dato risposte concrete agli studenti che vogliono, davvero pacificamente, risposte concrete. Ringrazio di nuovo il presidente Possa per la correttezza di quanto ha detto.

La ringrazio, Presidente,

in particolare, ve ne sono tre che sinteticamente cercherò di sottolineare. Il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame attiene al tema dell'autonomia universitaria, che viene stabilita sulla base della verifica di due presupposti: la stabilita la stabilita e sostenibilità del bilancio (che ha un contenuto chiaramente oggettivo) e i risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca.

nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Quindi, vi è chiaramente all'articolo 33 una riserva di legge allo Stato; sennonché il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, nel prevedere a forme di autonomia diverse da quelle previste in via generale, e collegando le stesse a queste due condizioni (ossia la stabilità prevista dal punto di vista del bilancio ma anche i risultati di elevato livello nel campo della didattica), affida

che queste possibilità di revisione dell'autonomia possono essere prese in considerazione e disciplinate con decreto ministeriale, in assenza di criteri predeterminati dalla legge. Ora, l'articolo 33 della Costituzione questo non lo consente: è necessario che vi sia una legge dello Stato che quanto meno indichi i criteri generali per poter intervenire in materia di autonomia. Affidare l'ampliamento o gli spazi dell'autonomia ad un decreto ministeriale è palesemente contrario all'ultimo comma dall'articolo 33 della Costituzione. inoltre, un secondo profilo di incostituzionalità. L'articolo 4 di questo disegno di legge afferisce ad un tema di grande importanza che è l'introduzione un Fondo per il merito volto a promuovere l'eccellenza e il merito tra gli studenti erogando premi di studio, buoni studio e finanziamenti. le modalità e la determinazione dei criteri di utilizzo del Fondo vengono affidati a decreti ministeriali di natura non regolamentare da adottarsi sentita la Conferenza Stato-Regioni. Senonché, la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 308 del 2004,

nonché le modalità dell'utilizzo del Fondo volto a promuovere l'eccellenza e il merito siano effettuate con decreto ministeriale sentita la Conferenza: è materia concorrente. Noi stiamo sottraendo, in violazione dell'articolo 117 della Costituzione, agli enti territoriali, alle Regioni, la possibilità di legiferare in questa materia. Non si può prevedere una consultazione, un parere; non si può fare con decreto ministeriale; non si può gestire questa materia con decreti ministeriali, perché è materia concorrente. Il terzo profilo riguarda Il terzo profilo riguarda alcune criticità sul modo di gestire la materia di questo provvedimento. Ne citerò una. Ci sono due materie estremamente simili che sono la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato e la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori

trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato - si prevede che la materia venga disciplinata da decreti legislativi, mentre nel secondo - revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori già in servizio - si prevede invece il ricorso a regolamenti di delegificazione. Su due materie analoghe non può prevedersi uno strumento normativo diverso: nel primo caso lo strumento è il decreto legislativo, nel

in riferimento alla determinazione di disciplina uguale, vi è una previsione di provvedimenti normativi diversi, e ciò va ad impattare con l'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, che ha individuato nel criterio di ragionevolezza anche uno degli elementi da prendere in considerazione nella verifica del rispetto del principio contenuto nel medesimo articolo 3. Nel momento in cui in questo provvedimento due situazioni giuridiche del tutto assimilabili vengono governate da provvedimenti normativi

a non procedere, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, all'esame del provvedimento che, così come è, su tre passaggi fondamentali (il trattamento del personale docente, la gestione del Fondo per i premi agli studenti meritevoli, l'autonomia universitaria), indubbiamente crea delle condizioni di incostituzionalità normativa tali da rendere questo provvedimento assolutamente fallace. Chiedo pertanto, ai sensi dell'articolo 93 del nostro Regolamento, che non si dia corso all'esame del provvedimento.

signor Ministro, colleghi, sono a chiedere di non procedere alla votazione del disegno di legge sull'università perché, sia in particolare per quanto riguarda l'articolo 33 della Costituzione sia per la sostanza effettiva del provvedimento, vi è il tradimento delle parole chiave con cui la stessa era stata presentata, parole chiave condivise anche dal nostro Gruppo, come autonomia, responsabilità, valutazione, merito, promozione del diritto allo studio. I provvedimenti adottati dal Governo in materia di università dimostrano come la politica dello stesso sul sistema di istruzione universitario non è finalizzata all'adozione di iniziative concrete per modernizzare le università, esaltando la loro autonomia finanziaria, introducendo forme sistematiche di valutazione efficace dell'utilizzo di risorse, incentivi e disincentivi, nonché aumentando la competizione tra gli atenei, ma al contrario si è realizzata e continua a realizzarsi in una serie di tagli che penalizzano l'intero sistema universitario. Le statistiche dimostrano che il nostro Paese è indietro rispetto alla media dei Paesi dell'Unione europea e dell'OCSE su molti parametri (numero dei laureati e dei ricercatori, investimenti per studenti, rapporto docenti-studenti). La percentuale del PIL destinata all'università è solo dello 0,8 per cento, a fronte di una media dell'1,3 degli altri Paesi. In particolare, il comma 2 dell'articolo 1, relativo ai principi ispiratori della riforma, prevede che «le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese diverse modalità di composizione e costituzione degli organi di governo». Tuttavia, tale maggiore autonomia è subordinata alla stipula di specifici accordi di programma con il Ministero. Tale previsione contrasta con l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, il quale dispone che le università «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato». La previsione dell'accordo di programma con il Ministero per sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi è indicativa di una volontà accentratrice, che di fatto mortifica e comprime l'autonomia degli atenei. Ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, i limiti dell'autonomia ordinamentale delle università possono essere stabiliti solo dalla legge. Il risultato di questa magnificata autonomia è di fatto il controllo degli atenei da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a sua volta sotto il controllo del Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 dispone che i regolamenti di delegificazione sono emanati nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge. Per la disciplina della materia, il disegno di legge fa un ampio e disinvolto rinvio, oltre che alla delega legislativa, a fonti secondarie, attraverso autorizzazioni alla delegificazione ed il rinvio a decreti ministeriali di natura non regolamentare. L'autorizzazione al ricorso a regolamenti di delegificazione per disciplinare il trattamento economico di professori e ricercatori, nonché la disciplina delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale si pone in contrasto con il principio della riserva assoluta nei confronti del potere legislativo, di cui all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione. Anche nel parere espresso dalla 1a Commissione del Senato, si evidenzia come la disciplina relativa alla valutazione dei candidati al ruolo di ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 2, «per il suo carattere di normativa di dettaglio, dovrebbe essere più opportunamente contenuta in disposizioni di rango secondario». Il ricorso a decreti ministeriali qualificati come non regolamentari appare un mezzo per eludere i vincoli normativi e procedimentali posti dalla legge n. 400 del 1988. Siamo dunque in presenza di un disegno di legge a dir poco inadeguato a far fronte ai gravi problemi dell'università, non dà alcuna risposta agli studenti e ai docenti e non introduce alcun progetto veramente innovativo, alcuna riforma dei meccanismi di ripartizione delle risorse, né tanto meno il rafforzamento dell'autonomia responsabile degli atenei. Infine, con questo provvedimento, si perde la straordinaria opportunità di varare una buona legge sull'università, che dovrebbe essere il luogo centrale della ricerca e dell'innovazione

Anche la Francia e gli Stati Uniti hanno aumentato i soldi per questo settore. I professori, i ricercatori e gli studenti che protestano pacificamente sono stufi di una classe politica italiana che non crede all'innovazione, che parla di sprechi ma attua tagli lineari. Il miliardo trovato all'ultima ora è una parziale e inadeguata restituzione del miliardo e mezzo di tagli operati dalla legge n. 133 del 2008 e prosegue una politica di risparmi fatta solo e soprattutto sul sapere e sulla conoscenza. È questo messaggio che il sapere, la cultura e la ricerca non producono che è sbagliato! Per tutti questi motivi, con un richiamo particolare all'articolo 33 della Costituzione, chiedo di non procedere alla discussione del testo,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1905-B. Il testo, infatti, definito dal ministro Gelmini una riforma epocale,

all'articolo 3 sul diritto di uguaglianza, all'articolo 117 sulle competenze delle Regioni, all'articolo 81 sulla copertura finanziaria. Contiene inoltre evidenti lesioni alle norme contenute nella legge di stabilità e nella legge di contabilità e finanza pubblica. Il testo appare poi con tutta evidenza più che una legge di carattere ordinamentale, più che una legge quadro che deve normare l'università, istituzione di alta formazione, decisiva per il futuro del nostro Paese, come un regolamento, fortemente centralistico, di estremo dettaglio e con numerosissimi rinvii a deleghe e ad altre norme di secondo grado.

L'articolo 29, comma 11, lettera *c)*, abroga il comma 11 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005,

è abrogato o è modificato? Penso che su questo passaggio ci sia una contraddizione che evidenza uno dei tanti errori e dei pressapochismi che sono contenuti nella elaborazione di questo testo di legge. Mi soffermo ora sugli aspetti di carattere costituzionale per segnalare molti elementi di incostituzionalità. Sottolineo, innanzitutto, la violazione totale del principio dell'autonomia universitaria, sancito dall'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione. A garanzia di questa autonomia, la Costituzione ha posto una assoluta riserva di legge per ogni normativa che si riferisca alla vita dell'università. È sufficiente considerare l'articolo 1 di questo disegno di legge per comprendere che si procede, invece, sull'aspetto organizzativo, sulla funzionalità, sugli aspetti statutari attraverso decreti del Ministro di natura non regolamentare. Pertanto, viene palesemente violata la riserva di legge, così come in un altro comma del medesimo articolo che prevede di procedere attraverso accordi Basta poi considerare il testo nel suo complesso per verificare che contiene normative di dettaglio, disposizioni che hanno più le caratteristiche di un regolamento e che sono assolutamente incompatibili con la valorizzazione dell'autonomia universitaria, disposizioni che, al contrario, sono poste in un'ottica centralistica e dirigistica. Come secondo aspetto, sottolineo la manifesta violazione delle competenze delle Regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, in materia di diritto allo studio e di istruzione. L'articolo 4 di questo disegno di legge norma il Fondo per il merito e rinvia alla definizione dei criteri per la gestione di tale Fondo a decreti ministeriali di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato‑Regioni. Sappiamo tutti che in materia concorrente, dove la competenza dello Stato concorre con quella della Regioni, lo Stato deve regolare tutta la materia con legge e non con dei decreti, tra l'altro di natura non regolamentare, e deve fare riferimento all'intesa con la Conferenza Stato‑Regioni, non al parere parere della Conferenza stessa. A dimostrazione della validità di quanto sto affermando, voglio richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 308 del 2004 che, con riferimento ad un fondo analogo, ha dichiarato l'incostituzionalità di tutte le norme riguardanti la gestione del fondo in quanto erano norme che davano tutto il potere decisionale agli organi dello Stato, ignorando la competenza delle Regioni. Allora mi rivolgo al ministro Calderoli, che è presente in Aula, e a tutti i componenti del Gruppo della Lega chiedendo loro se intendono mantenere un minimo di credibilità sulla loro politica presuntivamente federalista, se intendono dimostrare anche oggi che vogliono abbandonare totalmente questa politica o se, invece, pensano di potersi impegnare in emendamenti al testo proprio per correggere queste evidenti violazioni alle competenze e all'autonomia delle Regioni. Al ministro Calderoli, invece di fare improvvide dichiarazioni sullo spostamento dei Ministeri fuori da Roma, lo invito ad impegnarsi a ridurre e non ad aumentare, come avviene in questo testo, il potere del gigantesco, elefantiaco Ministero dell'istruzione; si impegni, accogliendo i nostri emendamenti, a riconoscere il ruolo che spetta alle Regioni.

L'articolo 4, comma 3, lettera *o)*, riserva una quota del 10 per cento delle borse di studio per merito agli studenti iscritti nelle università della Regione in cui risultano residenti. Innanzitutto, si tratta di un contenuto non condivisibile nel merito, in quanto è una norma che disincentiva non solo la mobilità sociale, come si registra in tutto il testo che stiamo discutendo, ma anche la mobilità geografica, contrapponendosi al principio che l'apprendimento si ottiene attraverso lo scambio culturale, attraverso lo scambio di esperienze, attraverso la mobilità degli studenti. Così come ci indica l'Europa, pensiamo ad esempio a tutti i numerosi progetti finanziati dall'Europa, quali l'Erasmus. l'Erasmus. Oltre alla non condivisione nel merito, c'è però una violazione evidente dell'articolo 3 della Costituzione, perché nulla garantisce che effettivamente vi sia il 10 per cento di studenti che ha le capacità e il merito per avere i premi di studio e che risiedono nella Regione in cui frequentano l'università. una lesione al principio di pari opportunità. Tutti questi aspetti sono stati già rilevati nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali del Senato, a cui rimando, perché vi è ancora un lungo elenco di articoli che vengono giudicati ai limiti della incostituzionalità e vengono evidenziati inoltre molti elementi di irragionevolezza. Da ultimo, faccio riferimento al tema della copertura finanziaria e al fatto che vi sono molte norme in questo disegno di legge che contrastano con la legge di contabilità e con l'articolo 81 della Costituzione, primo tra tutti l'articolo 4 che prevede premi, borse di studio ed altro senza avere alcuna previsione di copertura finanziaria, quando è del tutto evidente che, per fare un fondo, questa copertura deve assolutamente esserci. Del resto, questo articolo si colloca in un testo che nella sua complessità pretende di fare una riforma di carattere epocale non aumentando di un euro le risorse a disposizione, ma anzi tagliandone tante. Pertanto chiederei al Ministro che è qui presente, che è stato in Commissione con noi e ha parlato di queste risorse aggiuntive, e anche alla maggioranza di non ripetere in quest'Aula quanto effettivamente è stato detto tante volte, ossia che ci sono 800 milioni di euro aggiuntivi e che è necessario procedere rapidamente all'approvazione di questo testo perché questi 800 milioni debbono poter essere utilizzati. Credo che questa affermazione suoni davvero offensiva all'intelligenza di tanti docenti, rettori, studenti che stanno manifestando proprio per i tagli pesantissimi che l'università ha subito

gli 800 milioni previsti in aggiunta compensano solo limitatamente il taglio del fondo ordinario di funzionamento per l'università, perché nei fatti vengono tagliati 276 milioni.

questa volta lo facciamo in un momento ancor più difficile: la maggioranza, ormai sfiancata, giunta al capolinea, tira dritto, con la solita arroganza, a destrutturare l'istruzione pubblica e ad imporre questa indecente riforma universitaria, giunta faticosamente alla terza lettura presso quest'Aula del Senato. La posizione del Gruppo Italia dei Valori rispetto a questa riforma è stata ben chiara fin dall'inizio. Noi siamo fortemente convinti che questo modo di intervenire per riformare l'università sia assolutamente inadeguato e scorretto, essendo inimmaginabile pensare di riformare un settore così importante e così significativo senza un adeguato stanziamento di bilancio. Siamo ormai - e lo diciamo con grande forza - in piena emergenza democratica, sociale e culturale. Ormai è assolutamente chiara l'azione di questo Governo di considerare le politiche culturali, quelle legate alla scuola, all'università e alla ricerca, come marginali e secondarie rispetto alle politiche economiche e di bilancio. un testo approssimativo, signora Ministro, dalle conseguenze assai devastanti, che non soltanto inchioda gli atenei, ma determina, per l'intero mondo universitario, una pesante forma di estremismo burocratico. *(Brusìo).*

signor Presidente. Tale riforma - definiamola così - è finalizzata anch'essa a produrre indiscriminatamente risparmi al bilancio dello Stato e mortifica non soltanto la meritocrazia, ma anche l'autonomia, in un disegno preciso volto a realizzare un vero e proprio commissariamento delle strutture universitarie. Si tratta di un sistema paradossale, che vede le università sotto il controllo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e quest'ultimo sotto il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze. Complimenti davvero, signora Ministro! In tutto ciò, si segue sempre quello stesso copione che avete adottato per la scuola: operare tagli a non finire, senza alcuna considerazione nel merito, e poi dinanzi ai *media* negare tutto. È un modo davvero bizzarro di tranquillizzare la collettività! Quello che sconforta sempre più - e noi dell'Italia dei Valori lo abbiamo già detto e lo ribadiamo ancora una volta in questa occasione - è che emerge un quadro generale all'interno del quale non si capisce se lei, signora Ministro, sia consapevole di tutto questo o sia soltanto un mero strumento utile alla realizzazione di tali operazioni. Signora

risorse così limitate? Vorremmo capirlo, perché è la base di tutto. Avete concepito un'università pubblica di basso livello, a basso costo, e un'università privata di eccellenza solo per pochi. Siete riusciti anche ad ironizzare su tutti coloro che hanno posto in essere ogni forma di protesta, anche sui ricercatori che manifestavano sui tetti. Noi eravamo lì, con loro, insieme al nostro presidente Antonio Di Pietro. Pietro. Signora Ministro, quello era l'unico modo per far sentire la propria voce rispetto alla vostra arroganza e alla vostra inadeguatezza politica e culturale; quello era l'unico modo per cercare di stimolare forme di interlocuzione. Se vuole saperlo, noi staremo sempre dalla parte di chi vuol far sentire civilmente la propria voce. Non siamo solo noi dell'Italia dei Valori a chiedervi di fermarvi, ma è il Paese che lo chiede con forza: non potete restare sordi e ciechi dinanzi a tali richieste. Fermatevi! Siamo ancora in tempo. Tra l'altro, tale riforma vede favorite le università telematiche a danno dell'università pubblica. Ricorderà come tante volte, anche in sede di Commissione, tante volte, anche in sede di Commissione, abbiamo tentato di far comprendere le ragioni del nostro dissenso, anche suggerendo determinati correttivi, pur non condividendo affatto l'impostazione generale. Era un modo per cercare di limitare i danni. Tutto ciò purtroppo non è servito a nulla, neanche a limitare i danni, proprio per la vostra arroganza ed indifferenza! Non è superfluo ricordare che tra gli impegni altamente qualificanti di Lisbona 2010, assunti dagli Stati dell'Unione europea, vi era quello di attuare progressivamente politiche di bilancio che comunque dessero priorità all'alta formazione e alla ricerca pubblica degli Stati dell'Unione, atte a conseguire una destinazione di risorse nella misura non inferiore ad una percentuale del PIL di ciascuno Stato pari al 3 per cento. Nulla di fatto! stato pensato nella forte e convinta consapevolezza che l'Unione, la nuova grande realtà della politica mondiale, di portata storica, realizzata nel secolo scorso, dovesse puntare con determinazione ed assoluta priorità proprio sulle risorse inesauribili e sempre rinnovabili, seppure immateriali, del sapere, dell'intelligenza, della cultura, della fantasia e della creatività dei propri cittadini, specialmente delle generazioni più giovani. In tale contesto abbiamo più volte richiamato l'attenzione sulla necessità di garantire una sempre maggiore autonomia e professionalità delle istituzioni universitarie. Abbiamo richiamato l'attenzione, altresì, sulla necessità di concentrare sempre più risorse sufficienti per raggiungere e sviluppare l'eccellenza. Nello stesso contesto occorreva promuovere lo spazio europeo dell'istruzione superiore. Non le sfuggirà, signora Ministro, come in un contesto sempre più competitivo le università europee non potranno reggere i loro impegni istituzionali se non saranno messe nelle condizioni di operare al pari di quelle più moderne ed avanzate. Riqualificare le università e sostenerle economicamente nell'attività di ricerca dovrebbe essere l'impegno primario e preciso di ogni Governo. Ma voi siete molto lontani da questo modo di vedere. Se non si riconosce la priorità della ricerca e dell'istruzione, non si potrà mai assicurare al Paese un adeguato sviluppo. Noi siamo convinti che scuola, università e ricerca costituiscono, per definizione, il futuro delle nuove generazioni. Noi dell'Italia dei Valori siamo fortemente impegnati al fianco dei rettori, dei docenti, dei ricercatori, del personale amministrativo, di tutto il mondo universitario per fermare questo scempio. È a tal proposito che vogliamo differenziare le nostre posizioni, ribadendo che - a nostro avviso - il finanziamento alla ricerca non è un costo - come facciamo a farvelo capire? ma è l'investimento più alto e lungimirante che si possa fare per il futuro del Paese e delle nuove generazioni. È per questo motivo che cercheremo in tutti i modi di cancellare quello che avete fatto in questi anni. Cercheremo soprattutto di evitare, con tutti gli strumenti che il Parlamento ci consente, che l'Aula possa definitivamente approvare questa imbarazzante riforma. State scrivendo una brutta pagina della nostra storia, in danno della cultura e dei saperi. Assumetevi la responsabilità di tutto ciò. Noi non ci stiamo, e diciamo a gran voce no a questa riforma. *(Applausi

Onorevole Presidente, colleghe e colleghi del Senato, signora Ministro e signori del Governo, prendo la parola convinto che il disegno di legge che esaminiamo oggi in Senato, in seconda lettura, rappresenti un'occasione malamente gettata al vento dal Governo; l'occasione per ridare spinta a quanto è essenziale ad ogni società: produrre, trasmettere e diffondere conoscenza. In un Paese in grave ristagno, fortemente invecchiato, che arranca nei confronti internazionali, c'è un sistema universitario che ha urgente bisogno di una riforma con la R maiuscola, e non di una riformicchia, di un *bricolage* dell'esistente, come quella al nostro esame. Il ministro Tremonti, che si è assunto il compito di curatore fallimentare del sistema universitario, ha imposto il suo universale rimedio, che assomiglia a quello degli archiatri e dei cerusici di secoli lontani: salassare ripetutamente l'ammalato. Qualche pinta di sangue in meno non può che risanarlo, e questo mentre altri Paesi, con più intelligenza e ben maggiore lungimiranza del nostro, fanno la cura contraria, pur con Governi conservatori, come in Francia e in Germania.

Il secondo sta nel deprimere - invece di rafforzare - le capacità conoscitive, che sono l'insostituibile strumento per crescere e prosperare. Il terzo effetto è legato al secondo: chi consegue meno conoscenza è anche più vulnerabile e più debole. E così i risparmi di oggi in cultura e in istruzione si pagano domani in minore crescita e in maggiori spese per sostenere i più deboli. Meno istruzione, meno sviluppo e più *welfare:* è questa l'interpretazione della modernità dell'attuale maggioranza? Certo, l'università è ammalata. L'edificio ottocentesco che - bene o male - era stato funzionale alla società fino alla metà del secolo scorso, non ha retto ai ritmi dello sviluppo. Riparato, sopraelevato, ampliato, suddiviso, rabberciato, l'edificio è inadeguato alla democratizzazione e all'accelerazione del sapere. Molte sono le colpe di chi l'ha governato, dai professori ai presidi, ai rettori, ma anche dei Ministri e dei rappresentanti dei Ministeri che pur sedevano nei consigli di amministrazione degli atenei, anche di quelli che hanno sfiorato la bancarotta, L'università ha frammentato eccessivamente il sapere e le discipline, inseguendo acriticamente una domanda evanescente e poco informata; ha protetto le chiusure locali e disciplinari ed è in ritardo nelle aperture internazionali; ha scoraggiato la mobilità degli studenti e quella dei docenti; ha consentito che gli atenei si tramutassero in un lungo parcheggio per gli studenti, invece che in solerti officine di talenti; ha spesso preferito l'autoconservazione rispetto all'innovazione; troppo spesso è stata imboccata la strada della competizione con altri corsi d'insegnamento, con altri atenei,

pone l'Italia al settimo posto in campo internazionale; e ancora al settimo posto sta il nostro Paese nell'ambito della biologia molecolare e della genetica; un indicatore aggregato per le ma non siamo nemmeno tra i reietti; nella classifica scientifica abbiamo analoga posizione a quella che occupiamo nella classifica del PIL, o in quella - che fa gonfiare il petto di orgoglio a molti - dei medaglieri olimpici. Ora, dove e mai si fa la ricerca se non, quasi esclusivamente, nell'università? E da parte di ricercatori formati nell'università? E ancora, nell'ultimo decennio il sistema ha operato notevoli recuperi di efficienza: il personale è aumentato di poco, mentre il numero dei laureati è più che raddoppiato. Laureati e ricercatori si cimentano in campo internazionale - sicuramente persone selezionate - se la cavano assai bene e competono, spesso con vantaggio, con persone, altrettanto selezionate, provenienti da altri Paesi. Ma il Governo ha inflitto un salasso; un salasso coerente con l'atteggiamento punitivo che ha sottolineato e amplificato le colpe e ha passato sottosilenzio i meriti. meriti. Ricordo che la signora ministro Gelmini e il Presidente del Consiglio, qualche giorno prima dell'approvazione in prima lettura in Senato di questo disegno di legge, lo scorso luglio, mandarono un segnale tanto emblematico quanto inquietante alla comunità universitaria. Essi resero visita ufficiale al campus di una neonata pseudo-università telematica, l'unica che sia stata istituita (era ministro Letizia Moratti) nonostante il parere contrario del Consiglio universitario Un monumento non alla meritocrazia, invocata e sbandierata ad ogni passo, ma alla "somarocrazia" generata da pseudo-istituzioni di dubbia serietà, che il Governo sembra prediligere. Il disegno di legge torna al Senato dalla Camera dove ha subito un *maquillage* per lo più peggiorativo, anche se la sostanza rimane la stessa. Forse che questo provvedimento, riconoscendo la durezza dei tagli ai fondi pubblici, si preoccupa di porre le condizioni per attrarre i finanziamenti privati, con un'intelligente politica fiscale? Giammai, non avesse ad offendersi il Ministro dell'economia. Dà forse sostanza all'asserita ispirazione liberale del provvedimento, permettendo agli atenei di organizzarsi al meglio, seguendo la vocazione e l'opportunità? Non se ne parla nemmeno. Centralizza a tutto spiano e commissaria l'istituzione sotto un diluvio di norme e di prescrizioni, peraltro eludibili da accordi di programma di natura discrezionale. Incoraggia gli studenti che meritano? Solo a parole, con le medaglie di latta erogate dal Fondo per il merito, un salvadanaio senza denaro pubblico e con poca speranza - così come strutturato - di attrarre l'obolo privato. Si occupa del diritto allo studio? Ma quando mai! Ci pensino pure le Regioni, e che a meno dell'8 per cento dei meritevoli aventi diritto sia assegnata una borsa di studio e che meno della metà degli assegnatari ne fruisca, non interessa al Governo. Valuta il merito degli Atenei, dei dipartimenti, dei docenti della ricerca, degli studenti? A parole, perché l'ANVUR (l'agenzia di valutazione) è tuttora un guscio vuoto. Il suo sito ufficiale è composto di sole - ripeto - e imbarazzanti, pagine *web*. Gli organi devono ancora essere nominati. Eppure, per affrontare la mole di lavoro che la legge gli affida, l'ANVUR dovrebbe avere centinaia di esperti e di tecnici e dovrebbe già avere scaldato i motori. Offre la legge una soluzione al problema dell'invecchiamento del corpo accademico, dovuto alla mancanza di ingressi di giovani alla base della piramide? Non sembra proprio e in più pone quasi metà del corpo accademico - i ricercatori - su un binario che, se non proprio morto, è moribondo, per assenza di finanziamenti e di prospettive. Né, infine, il provvedimento ha avuto il coraggio di affrontare altri temi insidiosi, quale, ad esempio, quello di articolare l'ordinamento separando, con autonomie e responsabilità particolari, le facoltà professionalizzanti dal resto dell'università.

mi limito ad alcuni aspetti. La sfiducia nell'università e nelle capacità di chi la abita è tale, che il piano strategico dell'università - che significa soprattutto scienza e insegnamento - è approvato dal Consiglio di amministrazione, organo tecnico-gestionale, anziché dal Senato accademico, organo scientifico. Nell'organizzazione interna di ciascun ateneo rimangono assai confusi i rapporti tra dipartimenti, facoltà o scuole, e s'impongono numeri e limiti standard, precludendo agli atenei la potestà di articolarsi secondo logiche proprie, salvo a valutarne a posteriori il grado di successo conseguito.

C'è poi un concorso locale tra gli abilitati: il primo, la lista nazionale, sarà un filtro debolissimo; il secondo, una selezione influenzata dalle logiche locali, che accentuerà il provincialismo e le distanze tra atenei. Sul Fondo per il merito: quale privato vorrà mai mettere denaro nel fondo, organizzato secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e senza un soldo pubblico? Un privato che pagherà gli oneri gestionali del fondo, potendo far parte, tutt'al più, di un Comitato consultivo dei donatori? Cosa accadrà dell'attuale ruolo dei ricercatori - quattro docenti su dieci - la cui mobilità in ascesa è bloccata dalla regressione dei finanziamenti? Signor Presidente, c'è un consenso diffuso sulla necessità di valorizzare il merito, di adottare meccanismi di valutazione per farlo risaltare, di concedere autonomia, che implica assunzione di responsabilità. Ma questi principi, pur tanto sbandierati dalla maggioranza, sono traditi dal disegno di legge: non si valorizza il merito creando un fondo senza risorse e lesinando sul diritto allo studio, mentre si erogano fondi pubblici ad istituzioni private non di rado di dubbia reputazione. Meritocrazia o "somarocrazia"? Non si fa valutazione a parole, ma costruendo le capacità per farla e se l'ANVUR è un *mantra* evocato ad ogni passo, esso è anche un fantasma. L'autonomia poi, è costretta al guinzaglio dalle centinaia di norme e regole che la legge impone. Il Partito Democratico, che voterà convintamene contro questo disegno di legge, è pronto per una coraggiosa riforma, non per un *bricolage* dell'esistente. Due milioni di studenti, due milioni di famiglie, centomila persone che lavorano nelle università hanno diritto di chiedere di più e di meglio.

Assemblee parlamentari - la seconda in Senato - la discussione di uno dei più importanti provvedimenti di questa legislatura, che attiene ad un settore strategico per il Paese: la riforma dell'università. La scelta compiuta dal Governo ha incontrato, com'è noto, difficoltà di ordine economico dovute alla crisi globale che investe i processi di crescita, di sviluppo, di occupazione della nostra società occidentale. Ma si tratta di scelte e decisioni che finalmente faranno piazza pulita di finanziamenti a pioggia, indipendentemente dalle capacità di sviluppo e di produzione scientifica e culturale. Ed ancora: si tratta di scelte e decisioni che mirano all'eliminazione degli sprechi, all'abolizione dei corsi che hanno pochissimi iscritti e alla soppressione di quelle sedi distaccate che non producono assolutamente alcunché. La legge innova la *governance* delle università, immette personalità non accademiche nei consigli di amministrazione, limita a sei anni la durata in carica del rettore. Ma il vero perno della riforma è la valutazione degli atenei da parte dell'ANVUR, che anch'io anch'io auspico decolli quanto prima perché è fondamentale, cui sarà legata una quota importante dei finanziamenti statali, oltre a coniugare in maniera molto stretta l'autonomia con la responsabilità. Innumerevoli sono stati i tentativi di riforma dei nostri atenei lungo l'arco della nostra storia repubblicana. Ma ora, giunti al giro di boa del primo decennio del nuovo secolo, la crisi dell'università si caratterizza non più come la crisi di una semplice istituzione, ma di quello specifico e fondamentale organismo - l'università - che, formando la classe dirigente nei vari settori della medicina, della fisica, delle scienze economiche e giuridiche, della letteratura e della cultura, contribuisce e contribuirà sempre più al progresso del Paese.

Mentre in Commissione si era, pur nelle differenze di schieramento, ben lavorato, tanto che molti emendamenti dell'opposizione, lo voglio ricordare, erano stati accolti sia dal Governo che dalla maggioranza, in Aula si è preferito abbandonare completamente la ragione della riforma, in gran parte condivisa, e percorrere la solita strada dell'irresponsabilità, quasi nella consapevolezza che l'università non sia un bene di tutta la società; in parole povere, si doveva cavalcare la piazza. Del resto, come non confrontare i due testi di riforma, quello del Governo e quello del Partito Democratico, sottoscritto tra gli altri, lo vorrei ricordare, dalla senatrice Finocchiaro, dal senatore Zanda e dal senatore Latorre? Ma la domanda che spesso mi pongo e mi sono posto è se questi sottoscrittori così importanti del Partito Democratico abbiano o no letto il proprio disegno di legge. Credo che non lo abbiano letto. Ad esempio, oggi ci accusano di privatizzare le università perché nel consiglio di amministrazione, sulla base del testo del Governo, si apre timidamente all'esterno; vorrei ricordare che già adesso in molte università vi sono esterni, in quasi tutte. Ebbene, nel testo del Partito Democratico, al comma 7 dell'articolo 5, si afferma che almeno un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione è formato da esterni; e questa sarebbe la nostra privatizzazione? Potrei continuare con i poteri attribuiti al rettore e la durata della sua carica, con i poteri del consiglio di amministrazione e la durata del mandato dei suoi consiglieri (pensate, fino a otto anni; di più, con la possibilità di essere rinnovati per altri otto). Al rettore, pensate, viene attribuito il potere di nominare non solo la metà dei consiglieri ma anche di nominare il direttore generale, per cui verrebbe ad avere la maggioranza assoluta nel consiglio di amministrazione. Giustamente voi rispondete: «Sì, ma il consiglio di amministrazione può sfiduciare il rettore»; quando lui nomina la maggioranza assoluta? Questa purtroppo è la democrazia della sinistra. Tornando al disegno di legge del Governo, possiamo dire che si tratta di una riforma organica, che per la prima volta affronta i veri nodi dei nostri atenei: primo fra tutti il problema del reclutamento dei professori, nel contesto di una più generale riforma dei meccanismi di governo, di gestione e di organizzazione dell'istituto universitario. Nel corso dell'*iter* parlamentare ci siamo sforzati di trovare una soluzione ragionevole anche ad uno dei problemi più spinosi che avevamo ereditato: quello dei ricercatori di ruolo, i quali lamentano, a ragione, un ritardo trentennale della politica nel definire chiaramente la loro funzione e i loro compiti. Ma nei loro confronti c'erano da prendere delle decisioni,

oppure di rendere possibile un avanzamento di carriera basato sul merito, secondo regole stabilite dal disegno di legge. Si è scelto di andare in questa seconda direzione, fra l'altro apprezzata dalla maggior parte dei ricercatori, che chiedono di essere valutati per i propri meriti e di non venire accomunati in un provvedimento collettivo che ne svilirebbe il profilo scientifico.

tratta di professori di scuola superiore o di scuola media, ma di docenti universitari. La risposta a questa esigenza è stata di introdurre una chiara distinzione tra reclutamento e promozione. Per diventare associati od ordinari si deve conseguire un'abilitazione scientifica nazionale, che deve essere rigorosa e trasparente e che consente poi di partecipare a procedure rapide di selezione bandite da ciascuna sede. Ecco, direi che la forza del provvedimento sta proprio in questa organicità; nel senso che per la prima volta il Governo e il Parlamento hanno l'occasione di offrire al nostro sistema universitario un modello compiuto e coerente, non già disegnato sulla base di pregiudizi ideologici o su impianti organizzativi e gestionali di natura elefantiaca, quanto piuttosto su analisi ampiamente condivise dei problemi dell'università e maturato nella consapevolezza che è venuto il momento di dare risposte concrete ai problemi annosi dei nostri atenei: come quelli dell'autonomia - che non può essere anarchia, per cui ognuno fa quello che gli pare, come nelle pregiudiziali si paventava di una nuova programmazione dell'offerta formativa, di nuove politiche di diritto allo studio in una società che cambia e si trasforma, nonché di un reclutamento trasparente e meritocratico e di una diversa allocazione delle risorse. Questi sono i temi. E su questo il Governo e il Parlamento hanno lavorato. Su queste linee normative di fondo abbiamo voluto dare concrete risposte alle aspettative dei molti ricercatori che attendono di vedere riconosciuti i propri meriti. Oggi, signor Presidente, si è resa necessaria ed indispensabile una forte e pronta assunzione di responsabilità. Ed è la responsabilità e l'impegno che ci siamo assunti due anni fa e ci stiamo assumendo oggi, nel momento in cui ci accingiamo ad approvare definitivamente questo disegno di legge. Un provvedimento, ribadisco, davvero indispensabile se vogliamo dare un contributo concreto ad un processo di risanamento di cui già si intravedono i primi significativi segnali. Perché, onorevoli colleghi, in questi due anni che ci separano dall'avvio dell'*iter* legislativo della riforma, le nostre università non sono state ferme. Pur in un contesto difficile, hanno continuato a svolgere la loro insostituibile missione di insegnamento e di ricerca e, soprattutto, hanno avviato importanti azioni di risanamento, accorpando dipartimenti, eliminando alcuni corsi di laurea inutili e spesso senza studenti, chiudendo, infine, sedi decentrate insostenibili. Perciò, al di là del clima politico complicato che abbiamo di fronte, al di là delle divisioni e contrapposizioni fra maggioranza e opposizione, sono convinto che quest'Assemblea dimostri il suo apprezzamento per questo disegno di legge e il suo interessamento per i nostri atenei, anteponendo l'importanza di questa riforma per l'università ai legittimi interessi di parte. È con questi sentimenti, aspettative e preoccupazioni che il Governo e la sua maggioranza hanno vissuto in questi due anni la riforma che andiamo a votare. Ma voglio concludere questo intervento con le parole del professor Luca Ricolfi: «Noi universitari dovremmo smetterla di pensare che tutto dipenda dalle leggi e dai regolamenti: la qualità della riforma dipenderà anche dal modo in cui sapremo farla nostra e usarla per costruire una università più degna di un Paese civile». Paese civile». Personalmente condivido totalmente queste affermazioni e vorrei che anche questo Parlamento fosse, nelle sue diversità di opinioni, più degno di un Paese civile. La ringrazio e dico al Ministro: vada avanti. Il Paese ne ha bisogno.

signor Presidente. «Non siamo studenti fuori corso dei centri sociali, ma cittadini stanchi di vedere calpestato il nostro diritto ad un futuro. Il problema non è solo il disegno di legge Gelmini: il problema è che l'istruzione e la cultura dovrebbero e devono diventare una delle priorità fondamentali del prossimo Governo, di qualunque colore esso sia. Noi abbiamo il dovere e il diritto di fare in modo che questo accada. Vogliamo e pretendiamo un progetto di riforma partecipato e condiviso da tutte le parti sociali e politiche, che sia in grado di dare una prospettiva a noi giovani». Queste erano le parole scritte sul volantino con cui gli studenti dell'Università di Ferrara hanno motivato, non solo al mondo universitario ma all'intera città, l'occupazione della Facoltà di architettura in modo assolutamente pacifico. pacifico. Questi giovani uomini e queste giovani donne hanno voluto capire, hanno voluto incontrare le istituzioni, i parlamentari: lo hanno chiesto. Purtroppo, capire la distanza enorme tra le enunciazioni fatte dal ministro Gelmini e la verità del provvedimento ha creato in loro sconforto, delusione e rabbia. Si sono chiesti: con quali risorse si pensa di fare la riforma se non si sono neppure recuperate quelle tagliate a partire dalla manovra del 2008? È vero, sono stati recuperati 900 milioni, era stato un taglio di 1,3 miliardi. Il merito? Dov'è il merito, se non ci si preoccupa di assicurare a tutti la possibilità di accesso? Dov'è il merito, se l'utilizzo del fondo oggi non finanziato non tiene conto delle condizioni economico-sociali di partenza? Che senso ha poi sostenere chi frequenta l'università nelle regioni in cui vive? Che valore ha la mobilità e lo scambio di esperienze e di conoscenze? Quanto vale la qualità nel CEPU? Autonomia e responsabilità contro il centralismo e la burocrazia: ma come sono compatibili con le 500 norme ed i 1.000 regolamenti che sono necessari per dare gambe a questo provvedimento? Che senso ha l'incombenza del Ministero su ogni scelta strategica degli atenei? Queste sono solo alcune delle domande che si sono posti e che noi del Partito Democratico abbiamo posto a voi in questi mesi. A noi avete risposto respingendo parte degli emendamenti; a loro, a distanza di 20 giorni, non un cenno di considerazione. Ed oggi ci troviamo di nuovo in una città blindata, dove la distanza tra le istituzioni chiuse nel Palazzo e i cittadini è diventata anche fisicamente più ampia, dove la legittima richiesta di confronto sulle motivazioni all'insostenibile riduzione del diritto allo studio, alla mortificazione della ricerca, al dimezzamento dell'offerta formativa, all'inconsistenza dell'abusata parola merito, alla gratuita consegna della *governance* degli atenei ad un consiglio di amministrazione misto si è trasformata in tattica poliziesca. Ma la questione che loro pongono, di cui sono sommerse da mesi le pagine dei giornali, le trasmissioni televisive, ma soprattutto i pensieri e le discussioni delle famiglie, è ben più ampia del disegno di legge oggi in terza lettura al Senato. È la prospettiva della loro vita e del futuro del nostro Paese: il grande dramma del nostro tempo, un tempo nel quale si nasconde la polvere sotto il tappeto e si continua a fingere di non vedere che ormai è diventata una montagna. Non si è voluto agire per tempo ed ora l'unica strada che sembra essere rimasta è quella dell'autoritarismo. Si continua a tappare la bocca al pensiero non allineato. Niente di nuovo! Allo stesso modo sono state trattate le segnalazioni e le proposte del Partito Democratico. Sin dalla manovra del 2008 abbiamo denunciato la gravità della situazione, i tassi di disoccupazione dei giovani, i quali hanno pagato l'80 per cento delle perdite dei posti di lavoro causati dalla crisi economica, a lungo negata e che oggi sembra già superata; l'aumento del tasso di abbandono scolastico, a cui avete risposto abbassando di un anno l'obbligo; l'inadeguatezza del numero dei diplomati, che avete affrontato con una riduzione senza precedenti dell'offerta formativa, chiamando anche quella riforma. Provate ad andare nelle scuole superiori del nostro Paese a verificare il cambiamento. Vi diranno che l'unica cosa che è cambiata sono le classi, passate da 20-22 a 30 alunni. Le percentuali dei laureati che mettono l'Italia nell'era della conoscenza in posizioni inaccettabili, la perdita di competitività e di crescita e le vostre decisioni sono state quelle di azzerare le risorse della ricerca e dell'innovazione. La centralità della questione è stata costantemente evidenziata da proposte che sono confluite in un piano straordinario per le nuove generazioni, che abbiamo presentato anche nell'ultima finanziaria. L'atteggiamento del Governo e della maggioranza è stato sempre lo stesso, quello mostrato verso i cittadini, gli studenti, i ricercatori ed i docenti che manifestano. Un insopportabile e pericoloso paternalismo, che offusca le menti ed impedisce di cogliere un'occasione straordinaria, quella di recuperare alla politica ed alle istituzioni l'autorevolezza necessaria per costruire insieme ai cittadini un nuovo cammino per il Paese ed un futuro migliore per i nostri giovani.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministro, membri del Governo, mi pare che si consumi in quest'Aula, attorno ad un argomento sul quale c'è stato un lungo percorso e, perlomeno in prima lettura in parte condiviso, una sorta di rivincita dopo il voto di fiducia. Non si possono fare i bei discorsi sul bene comune e l'interesse generale del Paese e poi trascinare nel fango una riforma che, a detta di tutti coloro che l'hanno letta (perché molti non l'hanno fatto), presenta tanti aspetti positivi. Questo è male! Sembra che ora si preferisca alimentare lo scontro politico, perché divenga la giustificazione dello scontro di piazza. Certo, così non si fanno gli interessi di quei ragazzi che forse neanche sanno che la riforma dell'università è voluta anzitutto per dare un futuro migliore proprio a loro. Non nego che vi possano essere alcuni aspetti che si sarebbero potuti migliorare, e magari interverremo con apposite leggi ordinarie successivamente, ma ora il tempo per farlo non c'è più. Il Ministero dell'università ha elencato tre conseguenze gravissime se la riforma non venisse approvata ora. La prima è la scadenza, prevista per il 31 dicembre prossimo, per attivare i concorsi per professori ordinari e associati; la seconda è il blocco dei concorsi da ricercatore; la terza riguarda l'impossibilità di erogare i fondi (circa 118 milioni di euro) stanziati per gli scatti di stipendio legati al merito. Penso però che sia lo stato attuale dell'università italiana a consigliare una rapida approvazione di questa riforma. Se diamo un'occhiata a quello che succede nelle 77 università italiane, si chiarisce subito che quella di oggi è un'occasione storica, che la politica non può perdere. Non si tratta di enfatizzare alcuni problemi reali per giustificare riduzioni di corsi e di finanziamenti. Il fatto è che la ricerca universitaria è diventata a volte un *optional*. Ci sono troppi corsi di laurea, doppioni inutili che non danno sbocchi lavorativi ai laureati. Abbiamo, per esempio, più facoltà di veterinaria in Italia

non si sono mai registrate proteste studentesche come accade ora. Non si possono liquidare certe situazioni dicendo che si tratta di un facile luogo comune. So bene che ci sono docenti e facoltà che lavorano e meritano il nostro rispetto. Allora mi fermo qui, con la convinzione che per costoro la riforma sarà un atto di giustizia. Esaminiamo dunque l'asse portante di questo disegno di legge, cioè il principio di autonomia, enunciato con chiarezza all'articolo 1, un'autonomia che un'autonomia che si estrinseca anzitutto nei nuovi organismi di gestione dell'università, che vede l'introduzione del direttore generale, scelto dal consiglio di amministrazione, un organo che separa le responsabilità formative e di ricerca da quelle gestionali. Ma la cifra dell'autonomia è data dai piani triennali di sviluppo, che rappresentano un alto momento di politica universitaria, e non è affatto vero che si riducono ad un'attività burocratica sotto il controllo del Ministero dell'università. Sono programmi e progettualità strategiche, che dovranno fare delle singole università quel grande sistema nazionale integrato funzionale alle esigenze di un Paese moderno.

L'autonomia dell'università, così come concepita nella riforma che stiamo per approvare, è un tassello di quel mosaico che compone, insieme a federalismo e sussidiarietà, un sistema di *governance* poliarchico, garanzia democratica dell'unità e della distinzione del Paese. Altri aspetti della riforma meritano apprezzamento, a cominciare dalla presenza di un minor numero di organismi assembleari rispetto alla situazione attuale. Ciò consentirà di far uscire da situazioni di conflitto di interesse i responsabili delle università e, grazie anche alla presenza di membri esterni, si riuscirà a garantire l'effettuazione delle scelte necessarie nell'esercizio di funzioni che ora sono meglio delineate. Questa riforma argina le degenerazioni nepotistiche, mette in campo meccanismi per evitare o almeno rendere più difficile il servilismo di università, nate come faro di civiltà, libertà e progresso, ad interessi spesso poco nobili. Si introduce un sistema trasparente nella selezione del personale docente, col sistema dell'abilitazione nazionale di durata quadriennale, che avviene con meccanismi di esclusione che garantiscono certamente maggior serietà. Vengono valorizzati i dipartimenti; se ne è parlato poco nei dibattiti, anche sulla stampa, eppure essi diventano il centro propulsivo per la ricerca e la didattica, in quella definizione di funzioni cui prima accennavo. Nasce il Fondo per il merito ma, soprattutto, merito e qualità entrano come paradigmi per tutte le attività delle università italiane. È vero che le università subiscono riduzioni di risorse; tuttavia meno che altri comparti, proprio per la vitale importanza che si riconosce loro; riconosce loro; meno anche grazie agli 800 milioni di euro che sono tornati in finanziaria a favore del Fondo di finanziamento ordinario e ad altre fonti di finanziamento.

Auspico comunque che nei prossimi anni possa aumentare l'intervento pubblico, ma anche quello privato, a favore della ricerca e della formazione, da cui dipende la possibilità di mantenere la competitività del sistema Italia ed un ruolo propulsivo

la condizione dell'università italiana. Una collega che mi ha preceduto parlava di abitudine a nascondere la polvere sotto il tappeto. Direi che forse, sia C'era un Governo Andreotti; ministro della pubblica istruzione era diventato un uomo caro alla storia di quest'Aula, Giovanni Spadolini. Non sospettabile di alcun eccesso o abuso di riformismo, Spadolini, diventato ministro, nel 1979 sbloccò i concorsi a cattedra; concorsi a cattedra nell'università italiana non se ne facevano da undici anni. Ma quando mi riferisco alla polvere sotto il tappeto

e venne a sapere che alla facoltà di scienze politiche dell'università di Roma il suo collega Renzo De Felice, dopo molti episodi squadristici, aveva smesso di fare lezione per non provocare, per non suscitare tensioni nella libertà di insegnamento. Il suo collega Rosario Romeo aveva dovuto abbandonare l'università italiana e chiedere rifugio nella collina di Fiesole al prestigioso Istituto universitario europeo in formazione. Ciò nonostante Spadolini, conservatore ma non privo di un suo senso di responsabilità, convocò il rettore e il preside della facoltà di scienze politiche e gli chiese se non si poteva far nulla per rimuovere questa situazione. Se vi proponessi di venire a commemorare Aldo Moro nella sua facoltà, nella facoltà di scienze politiche, voi che direste? Con coraggio davvero accademico - l'aggettivo limita il sostantivo - i due colleghi dissero che bisognava parlarne con il Capo della Polizia, con il procuratore capo, con il Ministro dell'interno. Spadolini nella sua tenacia, in una università di Roma che sembrava del tutto "coventrizzata", riuscì ad andare a ricordare il collega Moro in quella occasione. Ma era sostanzialmente una università che aveva abdicato a se stessa. Paradossalmente una linfa di riaggiustamento venne dopo, negli anni '80, con quel provvedimento che inserì i professori associati, perché l'università era ancora ferma allo scontro del '68. C'era chi voleva il docente unico, c'erano *tazebao* che evocavano il popolo vietnamita, quello palestinese, l'alleanza gramsciana tra contadini e operai e il futuro degli assistenti universitari. Lo firmavano i figli dei baroni, tutti diventati baronissimi negli anni successivi. Da questo punto di vista la legge dell'80 rimosse quell'equivoco dell'incaricato stabilizzato, creò il ruolo degli associati e creò anche il ruolo dei ricercatori. Ma forse, con un eccesso di demagogia o di comprensibile cedimento ai rapporti di forza nelle piazze, il ruolo dei ricercatori, invece che un percorso, divenne a vita; arrivavano fino a 65 anni,

Ora la riforma sradica questa vergogna di un'università basata basata sulle tasse di tutti (a me non piace usare l'espressione «dei poveri e dei ricchi»). Ma, colleghi della sinistra, il ruolo dei ricercatori fino a 65 anni, di ex contrattisti, ex assegnisti o quello che erano, che non hanno fatto neanche una recensione,

stupidaggini che rivelano soltanto cinismo, sia negli *slogan*, sia negli argomenti. Se noi vogliamo la libera competizione nelle università per scegliere i migliori, un certo precariato è fisiologico. Se poi volete guardare a modelli anglosassoni, l'università statale e il posto fisso non esiste per nessuno. L'unica università statale negli Stati Uniti d'America è l'Accademia militare di West Point. Mi dispiace che invece le università non statali italiane (in una di esse mi onoro di aver insegnato per molti anni), di fronte al contributo dello Stato non guardino in faccia a nessuno; mecenatismo ce n'è pochissimo, sia nella meritoria tradizione liberale della "Bocconi",

nei prossimi giorni dalla piazza, sarebbe una vittoria della sinistra o non sarebbe, piuttosto, una vittoria di quei rettori che vorrebbero sfidare il 26° anno? È accaduto molte volte che in nome del sessantottismo si sia imposta la più proterva «congiura dei baroni» e lo dico anche per nomi a me molto cari: furono Moro e De Martino e la loro insensibilità

lei si prenda pure il posto del sessantatreenne professor Compagna, ma lo deve proteggere da qualsiasi «congiura dei baroni»,

In questi giorni stiamo drammaticamente misurando la distanza enorme che si è scavata tra il Paese reale e i palazzi della politica: così è da settimane che il Parlamento va a rilento per la lunga crisi politica di questi mesi e per di più è ridicolizzato, fino a sembrare un *suk* di deputati. La nostra economia arranca, priva com'è stata e com'è di un Governo in grado di guidarla in questa lunga a drammatica crisi. Il precariato e la disoccupazione corrono, investendo sempre più frequentemente queste nuove generazioni che abbiamo visto protestare nelle settimane passate, rivendicando spazi e voce. Nella folla delle manifestazioni di questi giorni ci sono stati atti e comportamenti teppistici e criminali, e lo abbiamo denunciato e condannato con forza. la loro stragrande parte, i giovani in piazza sono studenti che, a differenza di quello che sostiene il *Premier*, studiano; e proprio per questo impegno nello studio, non accettano questo provvedimento. Altri sono ricercatori, che, a differenza di quello che sostiene lei, onorevole Ministro, lavorano con passione e competenza. Reclamano voce, questi giovani, e non solo; protestano perché loro, ricercatori e studenti, il vero futuro dell'università e del Paese, sono stati totalmente esclusi dal percorso di discussione della riforma: cosa che peraltro segna emblematicamente la cifra democratica di questo Governo. Per giunta, sono stati persino accusati di difendere baronie e privilegi. Per questo, oggi, il mio discorso l'hanno scritto loro: 13 ricercatori e 30 studenti dell'ateneo fiorentino. Sono costretto a sintetizzare, e per questa ragione le ho chiesto di poter allegare il testo. «Siete oggi a votare» scrivono «questo disegno di legge contro il quale da mesi noi, studenti e ricercatori, ci opponiamo fermamente, cercando di farvi capire i motivi della nostra preoccupazione. Invano». Dietro la propaganda del merito, dell'inefficienza e degli sprechi, della "epocalità" della riforma contro cui, secondo voi, si scaglia solo chi ha da difendere degli interessi e dei privilegi, avete cancellato le nostre voci, ridicolizzato le nostre espressioni di protesta, creato un clima di tensione che ha contribuito a dar vita agli scontri dell'altro giorno, con pratiche che non ci appartengono, che rifiutiamo fermamente e che nulla hanno da offrire al nostro movimento di protesta. Non abbiamo avuto modo di dire la nostra su questa riforma, che non ha chiamato in causa le parti vive dell'università, coloro che davvero non hanno voglia né di difendere i privilegi né di mantenere lo *status quo*. Vogliamo un'università moderna, efficiente, accessibile, libera e di qualità, cui l'accesso sia garantito, come sancisce la Costituzione, ai più capaci e meritevoli, a prescindere dalle loro condizioni economiche di partenza. Un'università che sappia formare i cittadini e i lavoratori del domani, che sia pienamente inserita in una società moderna e aperta, che tragga talenti e cervelli, senza farli fuggire, che garantisca futuro e non precarietà. Questa riforma non fa niente di tutto questo. Per questo non ci piace, perché si basa su una politica di disinvestimento culturale e finanziario, che è ormai un tratto caratterizzante della destra italiana. Ne sono esempio i tanti provvedimenti succedutisi fino a quest'ultimo, in una linea costante di tagli, ridimensionamenti, impoverimenti: dalla chiusura automatica di tanti corsi di laurea fondamentali per lo sviluppo tecnologico, ai tagli al diritto allo studio, al fondo di finanziamento ordinario, a quello di intervento integrativo e per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, arrivando al blocco del *turn over* e alle restrizioni alla didattica, passando per la possibilità di trasformarsi in fondazioni di diritto privato. Ci avete detto per mesi e mesi che questa riforma sarebbe "anti‑baroni", in realtà, va verso la rifeudalizzazione del sistema universitario. La composizione delle commissioni di concorso è stata ristretta ai solo professori ordinari, i tagli agli stipendi, che sono maggiori per ricercatori e professori associati, sono quasi nulli per i baroni. legge non prevede una stabilizzazione in ruolo dei giovani prima dei 38‑40 anni, con un percorso di accesso al ruolo docente che oscilla tra i 12 e i 20 anni. Il diritto allo studio è poi la vittima ideologica di questo Governo: si tradiscono le aspettative di tutti coloro che volevano veder realizzare un vero sistema in grado di sostenere lo studente meritevole lungo la carriera scolastica e universitaria. «Predicare e non praticare» sembra essere il *leitmotiv* del Governo, che ci accusa di non proporre, senza darci modo di parlare; di difendere i baroni, senza far niente per smontarne il potere; di volere la conservazione, senza capire che i primi interessati ad una riforma dell'università siamo noi. Lanciamo al Governo ed alla politica una sfida, quella al confronto con noi, aperto e costruttivo, che parta dall'università e affronti i mali dell'Italia di oggi». Ecco, onorevoli colleghi, questo è quanto ci dicono gli studenti. Il Governo farebbe bene, almeno stavolta, in queste ore, a tenere conto ed aprire un dialogo serrato con loro. Se si vuole, se c'è la volontà politica, ancora si può fare.

a poco più di un anno dall'iniziale presentazione alle Camere, avvenuta il 25 novembre 2009, stiamo finalmente per tagliare un altro importante traguardo. L'approvazione di questa riforma, fortemente voluta e sostenuta in primo luogo dalla ministro Gelmini e poi dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene, segna un momento di grande importanza - io direi storico - per l'università italiana. Tale significatività è già racchiusa ed esplicata nel titolo di questo disegno di legge: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario». colleghi, credo non si possa fare a meno di definire con orgoglio come ambiziosa una riforma che si prefigge di incidere, con efficacia ed efficienza, sui gangli del sistema universitario, che da tanto, troppo tempo, richiedevano un intervento coraggioso al fine di eliminare storture sistemiche che ne inficiavano e ne inficiano in modo significativo la qualità. Come definire, se non storture, il proliferare illimitato ed indistinto dei corsi di laurea, spesso più utili a calmierare qualche, non sempre legittima, ambizione personale che non a rendere un servizio collettivo? Come definire il sistema di selezione dei docenti che, tra l'altro, ha generato in qualche ateneo l'assunzione di parenti e familiari con conseguente eliminazione del criterio del merito? Come denominare un sistema che ha consentito, in certe università, ad alcuni rettori di ricoprire l'incarico a vita o quasi? Metter mano per provare a modificare il sistema sta provocando reazioni a difesa dei privilegi, non solo da parte degli studenti, e ne parleremo, ma anche di parlamentari più o meno illustri che si arrampicano sui tetti o del governatore della Puglia che proprio ieri, in una trasmissione televisiva, dichiarava testualmente: «Disegno terribile di omicidio dell'istruzione pubblica». Non sarebbe stato forse meglio provare ad approvare una riforma condivisa piuttosto che fare e dichiarare tali sciocchezze? Eppure, di cose positive da sottolineare ce ne sono, a cominciare dai chiari riferimenti ai concetti di autonomia e responsabilità, valorizzazione del merito e combinazione di didattica e ricerca. significative, poi, le norme di *governance*: prima fra tutte, quella che prevede l'obbligo di adozione di un codice etico che sancisce i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove l'accettazione di doveri e responsabilità e detta regole di condotta, al fine di evitare ogni forma di discriminazione e di abuso e di regolare i casi di conflitto di interessi. Di particolare rilevanza è la previsione di incompatibilità fino al quarto grado di parentela per le assunzioni in ateneo. Sono fondamentali, poi, le norme che prevedono l'introduzione della figura del direttore generale, che sostituirà l'attuale direttore amministrativo e sarà un vero e proprio *manager* dell'ateneo, con tutti i benefìci che ne derivano in termini di professionalità della gestione. Altrettanto importante è la fissazione del limite per cui i rettori non potranno rimanere in carica per più di un mandato e, quindi, al massimo sei anni. Infine, altamente rilevante è la chiara distinzione tra le funzioni del senato accademico e il consiglio d'amministrazione: il primo, infatti, avrà il compito di avanzare proposte di carattere scientifico, mentre il secondo (che prevede la presenza di componenti esterni all'università scelti tra professionisti di «comprovata competenza in campo gestionale») delibera, tra le altre cose, sulle funzioni di indirizzo strategico, sulla programmazione finanziaria e del personale, nonché sulla sostenibilità finanziaria delle attività e sull'attivazione o soppressione di corsi e sedi. chiara, quindi, l'attribuzione di maggiori responsabilità in capo a questo organo, al fine di migliorare l'azione di governo dell'università e conseguire benefìci in termini di efficacia ed efficienza amministrativa. Per brevità, mi limiterò ad evidenziare solo qualche altra previsione normativa che ritengo significativa. sottolineo la fissazione di un limite temporale ai contratti: pur capendo, a livello teorico, le preoccupazioni da più parti espresse circa un rischio di aumento del precariato, ritengo però che il nuovo sistema determini situazioni di chiarezza fondate sul merito e risponda alla fondamentale esigenza di porre fine al fenomeno, tutto italiano, dei cosiddetti ricercatori a vita. Altra norma degna di menzione è la previsione, accanto alla borsa di studio a sostegno degli studenti a basso reddito, del fondo per il merito, costituito da risorse che vengono assegnate a prescindere dal reddito per gli studenti iscritti al primo anno di università, dopo il superamento di una prova a livello nazionale. Per ultima, ma non perché sia meno importante, citerò la norma che disciplina i concorsi per l'assegnazione delle cattedre. La riforma prevede l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale come condizione per l'accesso al ruolo di associato e di ordinario. La predisposizione di una lista a livello nazionale dei professori idonei viene effettuata da una commissione nazionale, sulla base di specifici parametri di qualità. Quest'ultimo concetto, insieme alla prospettiva nazionale, costituisce il significato importante e di novità della norma. Ribadisco quindi il mio giudizio estremamente positivo su questa riforma, evidenziandone l'incisività e soprattutto il coraggio innovativo in un settore così significativo e delicato per il Paese. Nel dire questo, però, non posso non sottolineare in maniera critica alcune forme di protesta, perlomeno "irrituali", e gli scontri che hanno contraddistinto e accompagnato taluni passaggi parlamentari di questo provvedimento. Pur essendo sacrosanto e irrinunciabile il diritto alla contestazione, ritengo essenziale ribadire che ciò deve avvenire nel rispetto delle regole, così come deve essere in ogni società democratica, e rimanere nell'alveo della legalità, senza mai scadere nella violenza, che invece determina sempre, a prescindere, la delegittimazione persino della più meritevole e giustificata delle azioni di protesta. Mi chiedo: ma sarà nel rispetto delle regole democratiche scendere in piazza con passamontagna e casco integrale? Ma sarà nel rispetto delle regole democratiche mettere a ferro e fuoco le città, tentando di assaltare anche i luoghi simbolo delle istituzioni? Ma sarà nel rispetto delle regole democratiche che uno studente riduca in frantumi un casco sulla testa di un altro studente, procurandogli trauma cranico ed altre gravi lesioni? Ancora: ma sarà nel rispetto delle regole democratiche che qualche magistrato, più o meno illuminato, rimandi a casa questi teppisti, senza fargli passare nemmeno un giorno in galera? Io credo di no, e penso che, nonostante tutto, stiamo approvando una buona riforma. Ministro, vada avanti: noi la sosterremo convintamente.

Onorevoli colleghi, nella serata del 18 dicembre scorso è improvvisamente scomparso, all'età di settant'anni, Tommaso Padoa-Schioppa, insigne economista e ministro dell'economia e delle finanze nella scorsa legislatura. Nato a Belluno nel 1940, dopo un brillante percorso di studi concluso con il *master* in economia al MIT di Boston, ricoprì prestigiosi incarichi di vertice nelle principali istituzioni italiane ed internazionali, in cui diede prova di straordinaria professionalità e preziosa dedizione all'interesse pubblico. È proprio con lo spirito di intelligente e leale servitore dello Stato che Padoa-Schioppa svolge prima il ruolo di responsabile della direzione generale degli affari economici e finanziari della Comunità europea, poi di vice direttore generale della Banca d'Italia e, successivamente, di presidente della CONSOB. Del suo stimato impegno professionale si ricorda in particolare il concreto contributo all'introduzione della moneta unica, nonché alla realizzazione e al consolidamento della Banca centrale e del sistema europeo di banche centrali. Ciò è testimoniato dapprima dall'intensa dall'intensa collaborazione con il presidente della commissione Delors e, successivamente, dall'incarico di componente del Comitato esecutivo della Banca centrale europea. Oltre a comprendere che il futuro del nostro Paese non avrebbe potuto prescindere dal rafforzamento della sua collocazione internazionale, ha avuto l'indiscutibile merito di evidenziare, sia nelle vesti di economista che di Ministro dell'economia, l'indispensabilità di politiche economiche dirette a contrastare l'insostenibile debito pubblico italiano. Tale visione, pienamente condivisibile, ha indubbiamente contributo ad attenuare per l'Italia gli effetti della recente crisi finanziaria internazionale. La Presidenza, nell'associarsi ai sensi di profondo cordoglio già manifestati ieri dal presidente Schifani alla famiglia del compianto professor Padoa-Schioppa, è certa di interpretare i sentimenti di tutti i colleghi nell'invitare l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio, in suo commosso ricordo. Consentitemi anche di aggiungere il mio personale cordoglio per un uomo di grande rigore, un economista autorevole e un convinto sostenitore della moneta unica europea. *(L'Assemblea

professor Tommaso Padoa‑Schioppa e il Ministro dell'economia e delle finanze del precedente Governo Prodi. Questi ricordi sono stati certamente adeguati alla sua preparazione, intelligenza, lungimiranza, al suo europeismo, che era assolutamente concreto e mai solo declamato, alla sua concezione delle istituzioni e del *munus* pubblico come bene raro in questa Italia confusa.

una limitazione provincialistica, perché l'Italia ha avuto e ha pochi uomini con questa straordinaria esperienza internazionale dei mercati, delle banche, della finanza e dell'economia del mondo. Molto è stato detto, e io penso di doverlo ricordare in quest'Aula, per fare una commemorazione che non sia soltanto rituale, affrettata e distratta Tommaso Padoa‑Schioppa uomo della politica perché è stato uomo di Governo: una dimensione sicuramente nuova nella sua esperienza professionale e umana.

in maniera determinante il ruolo, la funzione, le scelte e l'agire di Padoa-Schioppa come Ministro dell'economia e delle finanze di un Governo che - tutti lo ricordiamo - era chiamato a fare scelte assai difficili, che si sono rivelate assai utili per l'Italia

avemmo molti colloqui, alcuni per telefono, molti nel suo studio. Ricordo anche qualche pranzo di lavoro nella saletta dello stesso Ministero dell'economia.

nell'ascolto, perché la sua era la pazienza dell'intellettuale, che vuole capire fino in fondo un mondo, questioni, meccanismi, che gli sfuggono perché non li ha mai conosciuti, perché altra è stata la sua esperienza di lavoro, la sua esperienza professionale. Io ricordo queste lunghe conversazioni nelle quali mi invitava a descrivere minutamente i passaggi di ogni questione e aveva un'attenzione straordinaria anche alle sfumature degli argomenti e delle posizioni politiche che nel Gruppo e nella e nella maggioranza animavano la discussione. E questa pazienza dell'ascolto, questa umiltà di intellettuale nel cercare di comprendere non faceva poi nessun velo alla sua capacità di decidere ma era - io penso invece una caratteristica, una qualità del suo modo di esercitare le funzioni del governo, perché appunto la pazienza era uno strumento dell'intelligenza, della comprensione delle questioni. Certo, era una pazienza che portava alla decisione, e spesso quella decisione teneva conto delle argomentazioni che mi aveva chiesto di esporgli, ma aveva una qualità che troppo spesso - devo dirlo quelle discussioni non avevano avuto, cioè la lungimiranza. Non v'era una decisione che Tommaso Padoa-Schioppa non sapesse inserire in un percorso che andava oltre l'oggi, questa decisione in questo momento. E spesso diceva: perché oggi bisogna far questo, perché l'anno prossimo si potrà far quest'altro e poi ancora; esattamente la lungimiranza, la stessa lungimiranza che le cronache dei giornali di oggi ci hanno consegnato, la capacità di prevedere con così largo anticipo il fatto che il sistema finanziario mondiale avrebbe potuto soffrire di una crisi. E il tutto veniva fatto con con uno stile che non prevedeva né l'enfasi, né la retorica e neanche l'ombra della presunzione. Eppure diciamolo: avrebbe potuto benissimo permettersela; ne avrebbe avuto le ragioni. ma che si metteva a disposizione delle istituzioni, ovunque esse fossero, nazionali e internazionali, e del cambiamento e della sicurezza del vivere di milioni di persone, di intere economie. Proprio per queste ragioni io penso che quella di grande italiano sia una definizione appropriata. Ed è per queste ragioni che il mio Gruppo lo ricorda oggi con stima e con affetto.

ed era rientrato in Banca d'Italia. Ho visto per l'ultima volta sul piano personale Tommaso Padoa Schioppa venerdì della scorsa settimana, non questa ma quella precedente, a New York, ad un importante incontro in cui Tommaso ha svolto la sua grande ed efficace difesa dell'unione monetaria europea, dell'euro, della moneta unica, spiegando molto chiaramente quello è un passo fondamentale dell'Unione europea. Semmai c'è da discutere quale altra gamba affiancare alla stabilità monetaria e finanziaria, se la gamba della crescita, delle strategie per lo sviluppo di questo nostro vecchio continente. Quando si commemora una persona che ha percorso 30-40 anni, non solo in una singola disciplina, ma anche nell'impegno civile, è abbastanza ovvio che ci si riferisca a cosa pensava, a cosa ha prodotto e a cosa ha fatto. In questa memoria, anche per una piccola lezione collettiva, che è legata anche al tema che stiamo dibattendo in Aula (mi riferisco alla riforma universitaria), ricordare da dove veniva Padoa-Schioppa, da dove aveva costruito le fondamenta del suo lavoro scientifico e quindi capire che, a volte, le decisioni della politica producono grandi effetti positivi, ma possono produrre anche grandi effetti negativi, magari a distanza di dieci o venti anni.

sostenute da Luigi Einaudi e poi dai suoi successori, che mirava a fornire a parecchi giovani italiani la possibilità di avere solide radici e solide basi culturali di formazione scientifica, possibilmente all'estero. Questa cosa si chiama borsa di studio Bonaldo Stringher,

- quindi - come emigranti della prima ora bisognava andare in Inghilterra o negli Stati Uniti per fare il dottorato. Che frutto hanno dato Qual è il rendimento enorme per il Paese, oltre che per le singole persone, che ha prodotto quell'investimento in capitale umano fatto con tale lungimiranza, a partire - lo ripeto - dalle intuizioni, dopo la guerra, di Luigi Einaudi? di Luigi Einaudi? Ha prodotto una scuola e una formazione. Voi sapete quanto in quest'Aula, anche duramente, mi sono permesso di criticare l'amico Padoa-Schioppa, che era Ministro dell'economia, in un franco confronto di analisi e di proposte, ma in una filiera comune, che è quella di conoscere, prima di decidere; confrontarsi, prima di assumere decisioni. E questa non è una responsabilità che spetta soltanto alla politica: essa spetta all'intera classe dirigente, e certamente, *in primis,* alla politica.

professionale e scientifico di Tommaso Padoa-Schioppa nelle varie istituzioni, aveva messo alla base la conoscenza, costruendo per la prima volta in Italia, sul finire degli anni Sessanta e nei primi anni Settanta,

il confronto con quelli di altri Paesi. Si andava all'Università di Pennsylvania a confrontarsi, perché Modigliani dava una mano alla Banca d'Italia e alla Banca di Spagna a costruire il modello econometrico, ma lavorava con Ando alla UPenn per realizzare il modello econometrico della *Federal Reserve* (che poi si chiamò NPS). Questi mattoni di un percorso spiegano perché, come ha detto giustamente la collega Finocchiaro, nel ricordare Tommaso Padoa-Schioppa possiamo rammentare le sue idee, l'impegno civile e le posizioni che ha assunto, ma non possiamo dimenticare che, per ottenere questi risultati, oltre alla capacità della persona, occorre un senso di responsabilità collettivo nel sapere che le nostre scelte di oggi possono determinare (spero nel bene, ma qualche volta possono farlo anche nel male) effetti sulle future generazioni che che all'inizio, nei momenti in cui assumiamo delle decisioni, forse non percepiamo pienamente. Questo è il mio ricordo di Tommaso Padoa-Schioppa, anche se sul piano del confronto parlamentare, come ho già detto, abbiamo avuto modo di confrontarci anche duramente; peraltro, ho anche scritto un libro su quel periodo del Governo Prodi. È giusto, nel momento in cui si ricorda un amico, non far finta di non aver avuto divergenze, ma risalire alle radici comuni alle radici comuni che sono: conoscere, formarsi, riflettere e poi assumere le proprie decisioni o le proprie proposte politiche o di politica economica nella continuità intergenerazionale. Mi lasci citare solo un lavoro di Tommaso

contro la peggiore delle tasse, per far capire al sindacato italiano che l'inflazione e la rincorsa salari-prezzi era, prima di tutto, contro i lavoratori e il loro potere d'acquisto. Purtroppo, un altro amico, collega economista, è morto non in seguito a cause naturali, se pur tristemente improvvise come quelle di Tommaso Padoa-Schioppa: Ezio Tarantelli, morto per mano delle Brigate rosse per le sue idee.

fine che è la crescita e la prosperità in un collegamento tra le generazioni. La crescita non vuol dire solo proteggere la nostra generazione: vuol dire investire sulla nuova generazione,

ma creare nel nostro Paese le condizioni di lavoro e di interdipendenza con i grandi centri del mondo, in modo che la scelta se andare all'estero o restare in Italia sia una decisione personale e di opportunità. Oggi, purtroppo, questa scelta per i più bravi è a senso unico: i più bravi rischiano di dover andare e restare all'estero per avere opportunità di ricerca. Anche questo è il tema su cui dobbiamo riflettere in questo avvio di percorso

il mio Capogruppo, pochi minuti fa, ha affidato a me, che non sempre condivido le scelte dei banchieri, la commemorazione di Tommaso Padoa-Schioppa, stroncato nei giorni scorsi da un malore mentre era a cena in un ristorante romano in compagnia di amici. Come recitano le biografie, nasce a Belluno nel 1940, si laurea all'Università "Bocconi" nel 1966 e dal 1968, durante il movimento studentesco - quel movimento che voleva cambiare il mondo - inizia la sua collaborazione con la sede milanese della Banca d'Italia, raggiungendo il titolo di responsabile della Divisione mercati monetari del Dipartimento ricerca. Molti giornali ieri hanno titolato: «Un economista prestato alla politica, un guardiano dei conti con il vizio dell'Europa». È stato arcigno e severo: però, come ha ricordato la Capogruppo del Partito Democratico, Finocchiaro, è stato paziente, come sono pazienti i montanari, quelli che ascoltano gli altri in un momento in cui si cerca di non ascoltare le ragioni degli altri.

scrive: "Dal 1979 al 1983 Tommaso Padoa-Schioppa è direttore generale per gli affari economici e finanziari della Commissione delle Comunità europee a Bruxelles e inizia quindi il suo lungo e fertilissimo ruolo svolto nella costruzione europea un ruolo che già si delineava nei suoi esiti finali con il rilancio nel 1983 del progetto di una moneta unica europea. Uno dei padri dell'euro, insomma. "Si potrebbe proseguire ancora a lungo, ma forse non c'è bisogno. "L'unico rammarico" - scrive ancora il giornalista - "è la sua morte nel momento peggiore per l'Euro e per l'Europa. Chissà se la sua lezione servirà per costruirne una nuova". Muore proprio nel momento in cui

per la perdita di un europeista convinto, proprio nel momento di crisi, nel momento peggiore per l'unione monetaria (l'Europa delle monete non è l'Europa dei cittadini), nel momento in cui si vuole dividere, si porta l'attacco speculativo all'euro,

Noi, dell'Italia dei Valori, ricordiamo un europeista convinto. Non sempre siamo stati d'accordo con lui, ma proprio per questo tributiamo a lui e alla sua famiglia l'onore di un grande economista prestato alla politica.

al grande tecnico ed economista prestato alla politica e, se posso aggiungere, anche ad un amico con il quale ho condiviso una non piccola parte della mia vita politica. E il nostro pensiero, oggi, non può che andare alla sua famiglia e al grande dolore che sta provando. Vorrei perciò evitare, per quanto mi è possibile, di dare una lettura politica a questa commemorazione, ricordando in questa sede soprattutto le battaglie che ci hanno visto su fronti comuni e anche quelle sulle quali vi erano alcuni elementi di distanza, sempre peraltro possibili e, anzi, forse in qualche caso doverosi tra chi ha una visione puramente politica dei problemi e chi, invece, porta una convinzione e una visione soprattutto tecniche. Non si può non tributare un riconoscimento alto ad una persona che ci ha onorato, che ha onorato il nostro Paese, e che ha sempre svolto qualsiasi incarico abbia ricoperto, o sia stato chiamato a ricoprire anche lontano dal nostro Paese, con l'immutabile spirito di servitore dello Stato. Dal ruolo tecnico a quello politico, da quello europeo a quello nazionale e a quello internazionale, l'impegno di Padoa-Schioppa non ha mai guardato a interessi di parte ma unicamente all'interesse pubblico, andando spesso anche contro il coro di opportunismo politico senza il timore di alienarsi simpatie o facile consenso. Nel delicatissimo ruolo di Ministro dell'economia e delle finanze del Governo Prodi ha saputo distribuire, sempre con grande senso di responsabilità, i suoi sì e i suoi no ai Ministri e ai partiti che sostenevano quel Governo (e di questo io, pur se non facevo parte di quel Governo, sono anche un diretto testimone),

Quello che ha sempre saputo dimostrare Tommaso Padoa-Schioppa è una dote che non poteva non essere propria dell'uomo, prima che del politico, vale a dire la capacità di guardare avanti, di vedere le cose non solo nei dettagli ma in prospettiva. Possiamo definirlo certamente un uomo capace di visione, in un campo molto difficile, quello dell'economia e delle finanze, in cui, oltre alla capacità e all'intelligenza, bisogna avere delle doti non comuni per proiettarsi in un futuro, prossimo e anche più lontano. Non sembri strano oggi rivalutare alcune sue affermazioni, che sul momento potevano sembrare estemporanee e controproducenti. Mi viene da pensare a quanto aveva affermato in tema di "bamboccioni": un'espressione che al momento poteva sembrare urticante e ridicola ma che, rivista oggi con il senno di poi, può anche definirsi una previdente denuncia di una situazione che ogni giorno, sempre di più, si sta dimostrando una gabbia per lo sviluppo del nostro Paese, per il suo progresso e la sua crescita, poiché il blocco e la mancanza delle prospettive di futuro per i giovani sono sempre più spesso una costrizione e non una scelta. Come dicevo, non voglio dare una lettura politica, oggi, alla commemorazione di Tommaso Padoa-Schioppa. Voglio solo ricordarlo nei suoi caratteri distintivi, che non sono soltanto la capacità di proiettarsi nel futuro e di avere una visione, ma stanno anche nella capacità illuminata di leggere il presente e di trovare le soluzioni ai gravi problemi economici che noi soffriamo. la sua timidezza, la sua sobrietà ma, accanto a questo, la sua profonda determinazione, il suo rigore, una parola di cui spesso ci riempiamo la bocca e che, probabilmente, non sappiamo poi declinare al momento pratico. Voglio ricordarlo con il dolore per la perdita di una persona perbene, che credo resterà come esempio per noi tutti e per quella classe politica che proprio questa mattina, nel corso della trasmissione «Omnibus», ho inteso definire una classe politica che fa schifo. Credo che un giornalista ad «Omnibus*»* lo abbia detto, con profonda determinazione e convinzione. Questa non è una classe politica e tecnica che fa schifo. Quella che Tommaso Padoa-Schioppa ha rappresentato è la classe politica perbene che, lo voglio sperare, è la classe politica di tutti noi, di quelli che hanno a cuore il bene del Paese, l'interesse generale e che lo antepongono ai propri interessi personali.

sappiamo tutti come è andata); tale Documento conteneva addirittura, per rimanere all'attualità, la tabella con il rapporto docenti‑alunni, i confronti con i migliori Paesi europei e quello che si sarebbe dovuto fare anche in quel settore. Tommaso Padoa-Schioppa, o «TPS», come lo chiamavamo tutti per semplicità e anche con un certo affetto per la brava

La serietà e la concretezza dell'approccio, quel viso ieratico e lo sguardo fermo facevano capire fino a che punto egli comprendesse i problemi economici del nostro Paese. Da qui, anche il rigore spesso annunciato, che il Ministro all'epoca ha tentato di portare avanti, pur in una situazione complessa e fragile, spesso prendendosi colpe che non erano poi neanche tutte sue e critiche che non erano tutte rivolte solo

*(PdL)*. Signor Presidente, commemoriamo oggi un autentico *civil servant*, un economista autorevole e dotato di una straordinaria visione politica, quella più alta, espressa nelle istituzioni (e non solo) di cui orgogliosamente aveva fatto parte, come la Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione europea e la Banca centrale europea. Europeista assoluto, come altri hanno già ricordato, innamorato dell'idea spinelliana di un'Europa forte e gentile, capace di superare ogni ostacolo contrapposto dalla difesa, talvolta brutale, di interessi particolari definito giustamente l'«impeto intellettuale» e quindi padre fondatore della moneta unica: quella «moneta senza Stato», come diceva. A lui dobbiamo molto, proprio per quella lungimiranza che è già stata ricordata dalla presidente Finocchiaro. Egli stesso si definiva un keynesiano ma vero liberale, e in quella sintesi di profonde radici culturali e politiche si collocavano le sue più famose battute della sua breve carriera politica, che è stata ricordata dal collega Garavaglia qualche istante fa. Quella battuta molto famosa sui "bamboccioni" fotografava una generazione di giovani a cui va garantito un quadro normativo stimolante per la crescita della personalità e non solo indulgenza e comprensione. Chissà se è un caso che proprio oggi noi commemoriamo questa straordinaria figura di uomo intellettuale e politico mentre si discute dell'ultimo passaggio legislativo della riforma sull'università, in un clima avvelenato proprio da chi vorrebbe strumentalizzare quei giovani per scopi politici, fuori da quest'Aula, fuori dalle istituzioni, contro le istituzioni.

In Senato, il ministro Padoa-Schioppa aveva modo di difendere le sue scelte di Ministro citando Eraclito: «Combattere a difesa della legge è necessario per il popolo proprio come la difesa delle mura. Ritengo di avere combattuto a difesa della legge affinché la difesa delle mura continui a svolgersi nel modo migliore». Penso che citazione migliore di questa, in quella occasione ed in questa occasione, non ci possa essere per ricordare anche una sua famosa definizione, quella di "tesoretto", che lo rese famoso non solo ai *media* nazionali, ma a tutta la comunità intellettuale economica di questo Paese.

Bellissime forse non sono, ma certamente sono necessarie, e lui sapeva benissimo quanto fossero necessarie, perché sapeva riconoscere tra queste la tassa più ingiusta che tutti paghiamo, che era il costo, il peso di un debito pubblico tra i più alti del mondo. E proprio il suo rigore, quello che tutti noi qui oggi abbiamo ricordato, era ed è ancora ed è ancora per tutti noi, giovani e meno giovani, la migliore garanzia, la garanzia di continuare a dare stabilità al nostro Paese e una speranza al futuro di quei giovani che in molti vorrebbero difendere e che invece solo le istituzioni più illuminate, come quest'Aula, potranno difendere rispetto al loro futuro.

Signor Presidente, il Governo si associa alle parole di cordoglio espresse in quest'Aula dai rappresentanti dei diversi Gruppi parlamentari

svolto in modo del tutto disinteressato e lungimirante al solo servizio del Paese. Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, la politica deve essere sempre concreta, deve saper individuare, affrontare e risolvere i problemi partendo da principi chiari ed è questo ciò che cerca di fare il disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare. Uno dei difetti dell'università italiana è certamente la sua autoreferenzialità, un sistema di governo farraginoso che non favorisce la responsabilità delle scelte, un consiglio d'amministrazione e un senato accademico che oggi fanno le stesse cose, che sono espressione di corporazioni accademiche, sono strutturalmente inclini a scelte corporative. Si favorisce, in un simile contesto, una mediazione consociativa. Il sistema attuale vede una scarsa valorizzazione del merito degli studenti, una scarsissima valorizzazione del merito dei ricercatori e dei docenti. Con riferimento allo stato giuridico, devo dire che oggi vi è poca responsabilità: chi fa male il proprio lavoro, chi addirittura risulta assenteista non viene quasi mai sanzionato, non ci sono oggi i meccanismi adeguati per arrivare ad una sanzione. C'è, come dicevo, una scarsa valorizzazione di chi fa ricerca e didattica di qualità, è inesistente la differenziazione soprattutto per quanto riguarda le retribuzioni: che non si lavori o che si lavori non fa nessuna differenza. È difficile oggi persino la circolazione delle competenze: per fare un seminario in per fare un seminario in un'altra università è necessaria una autorizzazione e quindi occorre affrontare un percorso burocratico fastidioso. I finanziamenti devono essere legati sempre più alla valutazione dei risultati.

che induce a considerare soltanto le esigenze delle singole sedi, con una affievolita valutazione meritocratica di carattere più generale. Occorre

stimolando la produttività scientifica e finalizzandola alla carriera di professore. Va detto in questo contesto che la proposta iniziale del Governo conteneva anche numerose ombre, oltre a non dare,

la separazione netta fra consiglio di amministrazione e senato accademico; un consiglio di amministrazione aperto all'esterno, anche se è l'università che comunque decide sempre come aprirsi

Il senato accademico controlla l'operato del rettore e dello stesso consiglio d'amministrazione e può arrivare addirittura a sfiduciare il rettore. L'organizzazione interna degli atenei viene senz'altro semplificata, imperniata attorno al dipartimento, quale diventa la figura centrale e deve essere composto da almeno quaranta docenti. Il nucleo di valutazione ha poteri più incisivi per quanto riguarda anche i *curricula,* per esempio dei professori a contratto. Lo stato giuridico è senz'altro più liberale. Vengono finalmente e definitivamente introdotti scatti meritocratici al posto degli scatti automatici di stipendio. Si prevede un Fondo per il merito. Si favorisce la mobilità dei docenti e dei ricercatori. I finanziamenti sono legati alla valutazione dei risultati. È previsto l'accreditamento con un giudizio sulle singole università. È previsto il commissariamento delle università in stato di dissesto. Sono previsti interventi perequativi per le università sottofinanziate. È prevista l'abilitazione nazionale, ed è certamente questo un passaggio importante. È prevista una nuova disciplina degli assegni di ricerca, con una tutela previdenziale e una disciplina fiscale senz'altro più favorevole. Infine, si prevede la la contrattualizzazione dei ricercatori, ossia di quella posizione in ingresso che è tipica di quasi tutti gli ordinamenti a livello internazionale. Devo dire che alcune di queste linee, perlomeno quelle più contestate negli ultimi giorni, sono comuni anche alla proposta dell'opposizione. Se andiamo ad esaminare il disegno di legge presentato dal Partito Democratico, scopriamo curiosamente che

ai membri esterni, che sono esattamente un terzo dei membri esterni nel consiglio di amministrazione. Penso, per esempio, al ruolo del direttore generale.

e addirittura al modulo che viene lasciato indefinito di otto anni per il rettore, peraltro con possibilità di mandato unico.

anche alcune pecche: la istituzione della terza fascia docente e certamente un meccanismo molto più farraginoso di reclutamento locale conseguente all'abitazione nazionale, molto più complicato e certamente più burocratico. Ma è estremamente interessante che questo disegno di legge in qualche modo richiami svariate esperienze internazionali. Penso soltanto all'abitazione nazionale modellata sull'impianto francese francese e alla tanto contestata presenza di esterni che - si badi bene - non vengono imposti da presidenti di Regione o da associazioni di categoria,

Credo che, una volta fissati pochi paletti, come, ad esempio, quello del numero minimo degli appartenenti ai dipartimenti, forse era il caso di lasciare più autonomia. autonomia. Le scelte del Governo appaiono molto condizionate dal timore degli sprechi e ciò ha prodotto anche un eccesso di normazione, per cui alcuni commi probabilmente si potevano eliminare. Ma in un dibattito parlamentare così ampio, così complesso,

Il passaggio alla Camera non ha toccato punti essenziali del disegno di legge. Probabilmente lo ha peggiorato sotto il profilo della forma. Vi sono anche alcuni svarioni che magari potranno essere corretti in seguito, ma non intaccano la bontà complessiva del testo.

riferisco al ripristino degli scatti meritocratici che erano stati tagliati nella manovra di luglio. Dicemmo come fosse assai curioso che uno degli aspetti più significativi di questa riforma era propria l'introduzione di scatti non legati ad automatismi, ma ai risultati raggiunti dai ricercatori e professori e che la manovra di luglio aveva invece paradossalmente tagliato. Questi scatti sono stati ripristinati, così come è anche previsto un finanziamento della carriera per i ricercatori a tempo indeterminato, vale a dire la possibilità di assumere 4.500 professori associati, cioè cioè 4.500 persone che abbiano nel frattempo conseguito l'abilitazione ad associato. Non si tratta, dunque, di una *ope legis,* ma di un'opportunità concreta che si dà a coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione. La riforma si inserisce in un contesto di significative razionalizzazioni. Voglio solo ricordare che abbiamo ereditato un sistema in cui i corsi di laurea erano certamente ipertrofici a causa del tre più

Abbiamo anche ereditato un sistema in cui circa un terzo delle università aveva un rapporto tra fondo di finanziamento e spese per il personale del tutto al di fuori delle delle prescrizioni legislative. Anche da questo punto di vista, la legge inizia a fare chiarezza. Con la riforma, però, occorre iniziare a pensare al futuro dell'università italiana

una fase che necessariamente - su questo voglio essere chiaro sin da ora - non può prescindere da un incremento significativo di finanziamenti che invece

Parto da un argomento che di solito nelle nostre esposizioni arriva alla fine, perché, a ripensarci, mi sembra importante dargli il primo posto: la riforma costituisce una precisa lesione al diritto allo studio. Con il taglio delle borse di studio in realtà si interrompe una possibilità, come diceva la Costituzione, di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione della personalità umana.

Senza diritto allo studio non c'è diritto alla conoscenza. Si può studiare e non conoscere, ma il diritto allo studio dà accesso a questo diritto più alto, che in questa maniera viene invece negato. Si profila una condizione per cui si può temere un ritorno ad un rapporto tra studio e censo. Senza borse di studio, il censo rientra prepotentemente sulla scena. La troncatura del corpo docente, che sarebbe un argomento a parte e che cito solo di passaggio, rappresenta a sua volta una lesione del diritto allo studio, perché se si stabilisce un criterio per cui si ridurrà il corpo docente ad un quinto o ad un quarto e con metodi farraginosi, potrà sicuramente accadere che l'attesa di studio da parte degli studenti sarà diminuita.

rappresenta pur tuttavia il prodotto di una comunità scientifica. È fatto da persone che, anche se magari se ne sono allontanate, vengono da un'esperienza che ha consumato i problemi della ricerca e della didattica. Il consiglio di amministrazione è un organo che tiene fortemente alle ragioni di spesa. Consegnare le linee strategiche al consiglio di amministrazione significa rovesciare la logica, mettere il tavolo con le gambe per aria, come diceva un classico, instaurando probabilmente all'interno del Consiglio di amministrazione una logica che somiglia a quella del dominio lottizzato della politica. C'è chi ha parlato di consigli di amministrazione come ASL, dove è facile immaginarsi un processo lottizzatorio particolarmente non virtuoso. Un altro luogo comune di questa riforma è che finalmente inciderebbe sul potere dei baroni. Niente di più inverosimile, perché le commissioni di concorso sono attribuite

alla freschezza dell'indagine scientifica, cioè i ricercatori più giovani, le persone che sono ancora nel cuore, nel crogiuolo delle attività scientifiche, mentre spesso gli ordinari godono di una serena vecchiaia negli organi dirigenti. Questo rappresenta un danno specifico, perché è come se togliessimo alle commissioni di concorso l'occhio indagatore più efficace per individuare gli ingegni più promettenti. Scelte punitive per i ricercatori: argomento sul quale non mi tratterrò a lungo, e che è stato trattato da molti colleghi. Si determina una sorta di conflitto tra due tipi di ricercatori: i vecchi ricercatori sono condannati ad una sorta di evanescenza progressiva, mentre i giovani ricercatori sono sono infilati in un imbuto di precarietà che poi è selezionato da un processo di abilitazione nazionale che, come ha già detto molto bene il collega Livi Bacci, sul piano concreto non darà

Quando eravamo ragazzi e pensavamo a laurearci l'esempio cui si guardava sorridendo era quello di Piero Sraffa, vecchio amico di Gramsci, che era diventato celebre professore in Inghilterra scrivendo uno solo smilzo libretto, dal titolo strano: «Produzione di merci a mezzo di a mezzo di merci», che nessuno poi in realtà aveva letto e che veniva ammirato da tutti. Il professor Sraffa era diventato un grande autore con un libro solo. Quindi, la valutazione del merito è una questione delicata. Il problema è che tutto ciò messo insieme (il taglio del corpo docente, l'impossibilità della valutazione e il dominio dei consigli di amministrazione) determinerà sicuramente un impoverimento della ricerca, e l'impoverimento della ricerca determina un danno alla didattica. Vorrei concludere

è a proposito dell'impoverimento della ricerca. I tre professori piemontesi affermano che: «Comprimere la ricerca pura in nome di una qualsivoglia destinazione del sapere significa bloccarne la crescita. Scoperte e innovazioni sono possibili se si è aperti qualsiasi esito della ricerca, mentre esse sono fortemente inibite quando la finalità è è sempre già predeterminata dall'esigenza di un utilizzo economicamente e tecnicamente produttivo dei suo esiti». I professori citano un francese, Jean-François Lyotard, il quale scrive: «L'espansione della scienza non si produce attraverso il positivismo dell'efficienza. Al contrario: lavorare alla prova significa ricercare e "inventare" il contro-esempio, vale a dire ciò che è intelligibile; lavorare alla argomentazione significa ricercare il "paradosso" e legittimarlo attraverso nuove regole del gioco del ragionamento. In entrambi i casi l'efficienza non viene ricercata per se stessa: essa viene per eccesso, a volte tardi, quando quando i finanziatori si interessano finalmente al caso». Per concludere, voglio riferire anche una citazione che i tre professori piemontesi fanno di un celebre autore dell'idealismo tedesco, Schelling, il quale, nel 1841, in una sua prolusione all'anno accademico universitario affermava: «...da taluno vengono rimproverate le Università di tenere il giovane in uno stato di troppo grande astrazione rispetto al mondo (come se egli non esigesse proprio questo, che gli vengano garantiti in forma serena e non turbata lo sviluppo e la formazione delle sue capacità spirituali)...» - quasi il nostro dettato costituzionale - «proprio per questo» -aggiunge Schelling - «le nostre Università sono organismi ordinati, degni di essere mantenuti e degni di gloria». Nel 1841, a Berlino, si viveva sotto la monarchia assoluta prussiana: sembra che la monarchia assoluta prussiana fosse in grado di garantire il rispetto del'autonomia universitaria assai più della nostra democrazia. Signor Presidente, onorevole Ministro, il tormentato cammino di questa riforma evidenzia quante perplessità essa abbia suscitato dentro e fuori il Parlamento e come, quando si affronta un tema così complesso e così importante quale la formazione e la ricerca nel nostro Paese, ci siano ci siano molte questioni aperte, molte difficoltà e anche tante resistenze. È quindi evidente che consideriamo positivo il fatto che il Governo abbia immaginato di intervenire sul tema della riforma universitaria, ma temiamo che, all'esito di questo percorso parlamentare, questa riforma possa essere considerata un'occasione mancata. Non voglio qui fare il raffronto con tante altre riforme che sono state annunziate o approvate, i cui limiti però, nella loro pratica attuazione, riscontriamo quotidianamente. Fin dal primo momento, come Unione di Centro, abbiamo individuato la criticità di questa riforma, con riferimento, innanzitutto, al problema della sua

ciò che ci appare critico è che, più che trattarsi di una riforma che punti al rilancio dell'esistente e alla sua riorganizzazione in termini di efficienza, sia una riforma che punta al risparmio e che contiene in sé una serie di limiti che rischiano di determinare un arretramento rispetto al possibile sviluppo qualitativo delle università italiane quale asse dello sviluppo culturale ed economico di questo Paese.

soprattutto in questi frangenti, la risorsa più importante per un Paese come il nostro, che ha un grande patrimonio intellettuale e culturale, è investire nella ricerca e nella innovazione.

che ha tagliato al fondo di finanziamento ordinario risorse consistenti e tali da rendere insostenibile il sistema. Il Fondo con il quale oggi si coprono a malapena le spese del personale, ha subito con questo Governo una riduzione di 63,5 milioni di euro nel 2009, di 190 milioni di euro nel 2010, 316 milioni di euro nel 2011, di 417 milioni di euro per il 2012 e di 455 milioni di euro per il 2013: un taglio pluriennale che ammonta complessivamente a circa un miliardo e mezzo di euro in cinque anni. È vero che la legge di stabilità incrementa il fondo di 800 milioni per il 2011 e di 500 per il 2012, ma è una cifra inferiore a quella oggetto del taglio e crea un problema, visto che con queste risorse si devono finanziare anche, se non vado errato, i nuovi concorsi. In buona sostanza, il ministro Tremonti, che purtroppo ancora oggi rischia di essere il padre putativo di questa riforma, restituisce parte delle risorse sottratte al fondo ordinario, imponendo una riforma come condizione per recuperare soldi necessari al fine di evitare la crisi del sistema da lui stesso provocata. In realtà, dal punto di vista della criticità economico e finanziaria, il rischio di questo testo è che più che di un investimento si tratta di una vera e propria recessione. È, quindi, un'occasione persa - lo ribadiamo - perché siamo convinti che alcuni - e i più importanti - principi contenuti nel testo proposto e alcune soluzioni, anche obiettivamente innovative, siano utili e, anzi, indispensabili a correggere le distorsioni di un sistema universitario che si è radicato anche in corporazioni e privilegi, che non fanno onore fanno onore al mondo accademico e non aiutano gli studenti a migliorare le proprie condizioni di vita all'interno dell'università. Da questo punto di vista, signora Ministro, sono incerte le misure che consideriamo fondamentali per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, perché sono demandate a decreti delegati che non hanno una chiara copertura finanziaria. copertura finanziaria. Vi è un problema di compatibilità del testo rispetto alle previsioni dell'articolo 81 della Costituzione, laddove il disegno di legge, pur comportando una serie di oneri, non indica i mezzi per farvi fronte. Mi riferisco, in particolare modo, signora Ministro, all'articolo 5, commi 2 e 8, di legge dove si precisa che gli oneri derivanti dall'adozione dei decreti delegati, in considerazione della complessità della materia, non possono essere calcolati. Si riconosce, quindi, la possibilità che vi siano oneri, ma non si indicano i mezzi per farvi fronte demandando l'eventuale copertura ad altro provvedimento legislativo. Al di là della questione costituzionale, ciò che a noi preme in questo momento, proprio perché si tratta di un punto centrale di questa riforma, è che a questo testo e a questi decreti attuativi si dia compiuta attuazione in tempi rapidi, altrimenti anche il sistema su cui la riforma stessa si fonda rischia di non trovare alcun tipo di riscontro pratico e concreto. Sono invece certi i tempi entro i quali gli atenei devono rivedere gli statuti: sei mesi dall'entrata in vigore implementando un sistema organizzativo e gestionale analitico e rigido, uniforme per tutte le realtà, a prescindere dalle dimensioni e dalle caratteristiche;

poco razionali, laddove, avendo puntato su autonomia e responsabilità con allocazione delle risorse su base premiale, si dovrebbero lasciare gli atenei liberi di adottare il modello organizzativo che sia loro più congeniale. Saranno poi i risultati a decretare quali atenei sostenere economicamente per la qualità dell'offerta formativa e della ricerca e quali no. Questo secondo noi sarebbe stato un approccio molto più efficiente. efficiente. Ciò che viene configurato nel disegno di legge sembra più che altro una sorta di commissariamento preventivo, che può anche giustificarsi nella logica della deterrenza, ma che dal punto di vista funzionale e razionale sconta oggettivi limiti. Signora Ministro, riteniamo che questi siano i principali motivi di perplessità che hanno portato l'Unione di Centro e questo Gruppo a formulare diverse proposte che sono apparse come provocatorie, ma che in realtà sono funzionali a segnalare la circostanza che oggi è necessario un cambio radicale di rotta. Mi riferisco, ad esempio, alla proposta che abbiamo fatto sull'abolizione del valore legale del titolo per rendere veramente incisiva e certa la riforma, soprattutto nei suoi aspetti più innovativi. Concludendo, credo che una parola vada detta, e certamente né piacevole né positiva, sulla voce «diritto allo studio» a questioni che destano vivissime preoccupazioni. Il diritto allo studio è sancito dalla Costituzione, ma non sarà garantito perché, se da un lato, il disegno di legge introduce un apposito fondo nazionale per il merito, dall'altro non si definiscono i criteri di erogazione e, soprattutto, sono assenti i relativi fondi di copertura. Il reclutamento dei docenti, così come previsto, rischia di alimentare il precariato e di mortificare ulteriormente i giovani in quanto mancano le risorse finanziarie e quindi non ci sono garanzie sulle concrete opportunità di essere valutati ed inseriti. Non sono stati sufficientemente chiariti gli strumenti per i ricercatori in servizio e certo non può bastare la promessa di assumerne 1.500 per tre anni con i famosi 800 milioni, a fronte dei massicci pensionamenti e delle decine di migliaia il cui futuro è incerto a fronte del blocco del *turnover,* che certamente farà risparmiare al Governo ma non risolverà il depauperamento della didattica. Un'ultima considerazione, signora Ministro, riguarda l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario. È noto che è stata introdotta con un decreto-legge del 2006; in quell'occasione il Governo ha fatto ricorso ad un atto straordinario ed urgente per avviare l'Agenzia di valutazione. Ad oggi, però, questa Agenzia non ha in alcun modo operato questo aspetto, la valutazione, è strettamente collegato al senso, allo spirito alla finalità della riforma: mancando questo manca un pezzo importante. Se non si avvia il lavoro dell'ANVUR possiamo individuare nell'ambito del disegno di legge il comitato dei garanti e quant'altro ma alla fine tutto resta lettera morta e, sotto il profilo della parte più importante, cioè l'introduzione di parametri certi ed oggettivi per valutare la qualità del servizio universitario, non andiamo da nessuna parte. Per questa ragione abbiamo espresso ed esprimiamo forte critica per questo disegno di legge. proprio perché siamo innamorati del confronto parlamentare, che crediamo che sia la regola principale, e riteniamo che il merito delle questioni venga prima delle logiche di appartenenza e di schieramento, anche in questa sede, senza alcun ostruzionismo, abbiamo presentato pochi - otto - emendamenti ed ordini del giorno che segnalano le questioni politiche più importanti dal punto di vista del nostro Gruppo parlamentare. È quindi evidente che se nel corso del dibattito parlamentare su queste proposte politiche si dovesse registrare una convergenza da parte del Governo, non avremmo alcuna difficoltà a poter eventualmente anche cambiare il nostro orientamento di voto: ma sulle questioni vere e sui fatti e, soprattutto, sul percorso successivo di attuazione della riforma La riforma rinvia, con una serie di deleghe e di atti di natura regolamentare e non, a fasi successive in cui il Ministero diventa protagonista della concreta realizzazione dei principi che sono qui enunciati: è chiaro pertanto che noi siamo interessati a confrontarci anche sulla concreta attuazione della riforma e ci attendiamo che il Parlamento, anche su questo aspetto, possa dire con chiarezza che cosa si vuole fare e che il Governo e il Ministro ci dicano qualcosa

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, più di due anni fa siamo stati eletti con un solo scopo: fare le riforme per modernizzare il Paese. in quest'Aula per perseguire questo obiettivo e oggi siamo tenuti a confrontarci su un tema particolarmente rilevante e di comprovata essenzialità: la riforma universitaria. Il sistema universitario italiano ha una struttura che non premia il merito, non ci sono contatti con le imprese e gli atenei sono fabbriche di precari. La cosiddetta riforma Gelmini rappresenta un passo avanti, un distacco da questa situazione di staticità e di logoramento dell'istruzione; una riforma che ha l'intento di creare nuove basi per la formazione universitaria, che abbia come cardini meritocrazia e costi standard, affinché vi sia una redistribuzione equa delle risorse perequative sia agli atenei che agli studenti, in modo che vengano premiati coloro che sono più virtuosi. Inoltre, viene inserita l'incompatibilità tra parenti nelle assunzioni, soverchiando le logiche nepotiste della Prima Repubblica. Sulla riforma Gelmini è stata fatta tanta disinformazione, soprattutto per quel che concerne precariato e risorse disponibili. Ciò ha portato studenti - o presunti tali - ad occupare edifici e a salire sui tetti delle università: in questi giorni abbiamo assistito anche alla messa in scena di vere e proprie azioni di guerriglia da parte di delinquenti, falsi difensori della democrazia, che protestavano in nome del diritto allo studio e alla cultura. Ma la loro cultura civica dov'è? E' questo il futuro che vogliono? Un futuro fatto di violenza, picconi e bombe carta? Questa riforma ha come obiettivo la modernizzazione del sistema universitario in modo che si basi su una migliore formazione, sull'eliminazione degli sprechi e sulla creazione di una rete relazionale tra università, ricerca e imprese: essa vuole creare il futuro del nostro Paese. Questa riforma vuole fermare la fuga di cervelli. A dar manforte a questo mutamento è il progetto del Governo «Diritto al Futuro», che mette a disposizione 300 milioni di euro per lavoro e casa: un impegno segno di una particolare attenzione verso il mondo giovanile. Un altro esempio di questa attenzione è il prestito d'onore, prova tangibile dell'importanza che questo Governo ripone nella formazione quale base dei lavoratori di domani. La riforma Gelmini è l'ennesimo tassello del mosaico dell'operato di questo Governo del fare che ha ottenuto il mandato dagli elettori e che ha resistito anche alle congiure di palazzo, in nome del bene e del futuro del Paese. Riforma è sinonimo di innovazione e miglioramento: due sostantivi che incorporano perfettamente il senso e l'obiettivo del nostro programma di Governo.

Signora Presidente, come è ormai chiaro, il nostro giudizio su questo testo è molto negativo. Ed è negativo per una ragione semplice: perché non è all'altezza dei cambiamenti necessari, perché non risponde ai bisogni reali dell'università, perché l'università non è concepita come una delle molle dello sviluppo del nostro Paese. Il testo che ci ha restituito la Camera dei deputati è, se possibile, ancora più insoddisfacente di quello licenziato dal Senato in prima lettura. È più farraginoso, meno meritocratico, appesantito da procedure burocratiche, elefantiaco: nel disegno di legge e altrettante a venire nei decreti legislativi. Noi abbiamo riconosciuto che la discussione svolta in Commissione al Senato aveva apportato qualche modifica positiva al testo proposto dal Governo, nel quale fra le missioni principali dell'università mancava perfino la ricerca. Ma ora abbiamo un testo pasticciato, ancora pieno di centralismo, scarsamente rispettoso dell'autonomia dell'università. Se devo rispondere alla domanda sul perché di tanto accanimento burocratico, direi che è sbagliato il punto di partenza. Voi siete partiti dal presupposto che l'università sia un concentrato di baronie da punire, di poteri illegittimi da sconfiggere, e da sconfiggere ripristinando un anacronistico e arcaico centralismo, con norme eccessivamente e minuziosamente prescrittive. Il risultato sarebbe stato certamente più qualificante se si fosse partiti, come noi abbiamo proposto, dalle eccellenze di cui le nostre università, ancora, nonostante tutto, dispongono; se l'intento fosse stato non la punizione di docenti e rettori, ma la valorizzazione di ciò che va salvaguardato, la promozione dell'autonomia nella responsabilità, la qualità della didattica, il diritto allo studio: in una parola, se ci fosse stato investimento e non disinvestimento, con la conseguente riduzione delle risorse. Il risultato sarebbe stato diverso se la riforma fosse stata concepita come un'occasione per contribuire a costruire un'Italia più dinamica, più competitiva, più capace di cooperare a quel progetto tanto ambizioso quanto ineludibile di costruire un'Europa della conoscenza, un'economia fondata sul sapere, sulla ricerca. È stata per noi un'occasione persa; da voi è stata persa, perché questo Governo e questa maggioranza evidentemente credono poco a quel progetto e attribuiscono all'università e alla ricerca un ruolo marginale. Si tratta di un progetto forse troppo lungimirante per chi ha scelto di navigare a vista, nell'economia come in altri settori. Io voglio indicare alcune, soltanto alcune, delle maggiori criticità che ci portano a contrastare questo provvedimento. La prima criticità l'attacco all'autonomia delle università, che è un principio costituzionale. Autonomia e responsabilità avrebbero dovuto costituire il principio cardine di ogni riforma sulla *governance*. E, invece, in questo testo c'è poca autonomia e poca responsabilità. Alla responsabilità si può arrivare solo con una valutazione attenta dei risultati, con la premialità. Nella pratica dell'autonomia servono poche regole e molta sostanza. Signora Presidente, in questo modo non riesco a parlare, non riesco a concentrarmi. La qualità si esalta anche attraverso la differenziazione La qualità si esalta anche attraverso la differenziazione e la specializzazione; è l'uniformità che porta invece all'appiattimento. In questo testo così prescrittivo si ritrovano soprattutto lacci e lacciuoli che mortificano l'autonomia e rendono difficile l'esercizio della responsabilità. Anche le parti che riguardano la valutazione si perdono nel *mare magnum* di norme prescrittive e centralistiche. La seconda criticità riguarda il diritto allo studio la finta meritocrazia. Parliamo di finta meritocrazia perché non si può parlare di merito senza costruire pari opportunità. Noi siamo a favore della valorizzazione del merito, perché una società basata sul merito è più giusta, ma non c'è meritocrazia se non si è in grado di valorizzare i talenti, ovunque siano, a prescindere dalla provenienza sociale e familiare. Ciò che ad oggi abbiamo visto nella legge di stabilità è la riduzione delle borse di studio, che ha giustamente allarmato gli studenti, le famiglie e le Regioni.

perché non distingue fra abbienti e non abbienti, perché riguarda chi è già iscritto all'università, e dunque perché finirà per avvantaggiare chi gode già di vantaggi familiari e provenienza sociale. Non modificherà in niente la scarsissima mobilità sociale, e questo sì che favorisce e restaura il privilegio sociale. C'è poi un'aggiunta apportata dalla Camera all'articolo in virtù della quale si premiano gli studenti che frequentano l'università nella propria Regione. È chiaramente una concessione al localismo gretto della Lega, ma noi sappiamo che, riducendo la mobilità necessaria per andare a cercare le università migliori, si introduce un'ennesima penalizzazione dei giovani più meritevoli e bisognosi di essere sostenuti; si introduce il principio della discriminazione territoriale e si dà un colpo alla qualità. questa norma basterebbe a motivare il nostro voto negativo nei confronti dell'intera legge. Terza criticità. Si parla di merito e di qualità, ma poi troviamo riconoscimenti alle università telematiche: sarà una marchetta al CEPU, ben rappresentato in Parlamento e tanto affettuosamente trattato dal Presidente del Consiglio, come se fosse l'Università riconoscimento di crediti formativi ai vincitori di medaglie olimpioniche, quale che sia la facoltà frequentata. Troviamo poi delle assurdità, come quella di stabilire per legge un limite massimo e un limite minimo di pubblicazioni nelle procedure di idoneità: minimo dodici, si dice, indipendentemente dal settore disciplinare. In questo modo, la ricerca si misura a peso e non per qualità, che può essere rintracciata anche in poche pubblicazioni, come sa chiunque faccia ricerca. Inoltre, si pone il problema enorme delle risorse. Ormai l'hanno capito tutti che non ci sono risorse per la riforma: gli 800 milioni previsti dalla legge di stabilità sono solo un reintegro parziale di decurtazioni fatte in precedenti provvedimenti economici e rispetto al dovuto nel 2011. Di fronte alle contestazioni di studenti, docenti ed anche di rettori, la ministra Gelmini ha lanciato un assurdo e inaccettabile ricatto: non ci sono risorse senza riforma. Non si fa così, ministra Gelmini.

per rinviare alle calende greche nuovi ingressi nelle università. Noi dunque siamo contrari, perché questa specie di riforma blocca ed ingessa le università, perché penalizza i giovani nello studio, nella ricerca e nel dottorato. Non vi sono certezze per i giovani precari che già sono dentro, che meritano di restarci, perché di loro l'università avrebbe bisogno, ma che non trovano sbocco. Il reclutamento è bloccato: non si intravedono possibilità di reale dinamismo, mobilità, innovazione nel reclutamento; rimangono tante figure precarie. Ci sarebbe ancora il tempo per cambiare, per fare una riforma utile e innovativa. Voi questo lo state rifiutando. Avete fretta di arrivare, ma a danno della parte migliore dell'università e dei giovani, doppiamente penalizzati: penalizzati come studenti, sul piano del diritto allo studio che si riduce, come ricercatori che aspirano a qualche certezza per il loro futuro, sempre più precario. Se studenti e ricercatori protestano pacificamente non sarà perché non hanno capito, come qualcuno ha detto, ma perché hanno capito fin troppo bene che è in gioco il loro futuro.

il provvedimento alla nostra attenzione, che confido diventerà legge dello Stato entro pochissimi giorni, attua una coraggiosa e profonda modernizzazione del nostro sistema universitario, modernizzazione ormai assolutamente indispensabile per competere con successo nel sempre più difficile confronto internazionale delle economie. Il testo approvato dal Senato lo scorso luglio è stato modificato dalla Camera dei deputati essenzialmente con integrazioni. Sono stati aggiunti quattro articoli. Apprezzo vivamente l'inserimento nel provvedimento dell'articolo 19 («Disposizioni in materia di dottorato di ricerca»), che rafforza in modo rilevante la qualità e la serietà del terzo livello di laurea. Circa l'articolo 17, che stabilisce l'equipollenza con la laurea triennale dei diplomi rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali, purché conseguiti dopo un corso di tre anni, mi pare opportuna, signora Ministro, l'estensione a queste scuole di regolamentazioni analoghe a quelle stabilite per le università, onde promuovere e garantire anche in esse qualità e merito. Di assai minore rilievo e forse anche un po' opinabili sono gli altri due nuovi articoli: l'articolo 21 («Comitato nazionale dei garanti per la ricerca») e l'articolo 28 («Istituzione di un Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»). Nei 25 articoli a suo tempo approvati dal Senato la Camera ha aggiunto 28 commi. I più importanti sono gli 11 nuovi commi inseriti nell'ultimo articolo, l'attuale articolo 29 («Norme transitorie e finali»). In sostanza l'impianto del provvedimento è rimasto quello esaminato e votato al Senato. A questo punto può essere utile una breve sintesi degli elementi portanti del sistema universitario toccati e riformati dal provvedimento. Il quadro complessivo delle riforme dirette e delle riforme che verranno approntate nei prossimi due o tre anni (tramite decreti legislativi, decreti ministeriali, decreti interministeriali, regolamenti ministeriali, statuti universitari, regolamenti universitari, e così via) è impressionante. Il provvedimento, in particolare, al fine di determinare modalità di gestione più attente alle compatibilità di bilancio e alle esigenze degli studenti, prescrive l'adozione negli statuti delle università di una nuova struttura di *governance*, ridisegnando competenze, ruolo e procedure di nomina ed elezione, relative a rettore, Senato accademico, e Consiglio di amministrazione. Obbliga le università all'adozione di un sistema di contabilità analitica economico-patrimoniale, nonché a formulare bilancio di previsione e rendiconto secondo schemi di bilancio prestabiliti. Attribuisce ai dipartimenti (e non più alle facoltà) il ruolo centrale della struttura organizzativa dell'università. Modifica in senso nettamente meritocratico le modalità di distribuzione del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Definisce in dettaglio lo stato giuridico dei professori e degli attuali ricercatori a tempo indeterminato, prevedendo impegni vincolanti per didattica, in Consente d'ora in poi esclusivamente l'assunzione di ricercatori a tempo determinato (per un tempo massimo di 6 anni), individuando nel contempo per i ricercatori meritevoli un ragionevole percorso di accesso al posto di professore associato. Introduce valutazioni periodiche dell'attività di ricerca e della didattica dei professori ordinari e associati (fino ad ora poco o nulla sottoposti a valutazione). Stabilisce modalità di accreditamento e valutazione delle intere università. Innova profondamente le modalità di reclutamento dei professori, che saranno basate sul nuovo istituto dell'abilitazione scientifica nazionale (e sulla chiamata diretta degli abilitati da parte dei dipartimenti).

Riduce da sessanta a dodici il numero massimo dei crediti formativi che una università può riconoscere in base alle effettive competenze di uno studente. Revisiona la normativa di principio in materia di diritto allo studio, prevedendo la definizione, d'accordo con le Regioni, dei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle università statali, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore. Promuove l'eccellenza e il merito tra gli studenti, anche mediante un apposito fondo per il merito. Le varie centinaia di disposizioni contenute nel provvedimento, che determinano tale complessa e profonda riforma, sono tutte tese ad una comune fondamentale finalità, quella dell'elevazione della qualità delle università, qualità dell'insegnamento, qualità della ricerca, qualità dell'assistenza agli studenti. Fa veramente dispiacere riscontrare che il provvedimento, giudicato positivamente da molti autorevoli commentatori e addetti ai lavori, giudicato positivamente dalla stessa associazione CRUI di rappresentanza dei rettori delle università italiane, sia invece stato fortemente osteggiato dall'opposizione, sia in sede politica, sia nelle piazze. Questa durissima opposizione ha ritenuto - come abbiamo sentito anche adesso - che, nel loro complesso, le disposizioni del provvedimento riguardanti la *governance* delle università, e in particolare l'assegnazione al consiglio di amministrazione di un ruolo molto importante nella gestione degli atenei, costituiscano un grave *vulnus* all'autonomia universitaria tutelata dall'articolo 33 della Costituzione. Ha ritenuto che la partecipazione al consiglio di amministrazione di almeno 2 consiglieri non appartenenti all'ateneo (e almeno 3 nel caso più frequente di consiglio di amministrazione con 11 componenti) costituisca un rischioso e anche irresponsabile affidamento della gestione dell'università a chi può non conoscere affatto le sue delicate delicate funzioni di formazione e possa altresì essere prodromico a forme di parziale privatizzazione delle università statali. Ha insinuato senza alcuna giustificazione che l'apertura anche alle università telematiche dell'accesso agli incentivi per le università non statali legalmente riconosciute (di cui all'articolo 12 del provvedimento), preluda all'indebito favoreggiamento di una ben determinata università. Non ha espresso alcun apprezzamento riguardo a varie importanti disposizioni contenute nel provvedimento, che nel passato la sinistra aveva sempre sostenuto, come come - ad esempio - l'ampio riconoscimento del ruolo degli studenti nel funzionamento dell'università, la centralità del dipartimento nell'organizzazione della vita dell'università,

tende a ledere fondamentali esigenze di riequilibrio territoriale del sistema universitario del Paese. Ha criticato vivamente l'istituzione del fondo per il merito di cui all'articolo 4, ritenendola non allineata con le prioritarie esigenze di diritto allo studio. Ha sovrapposto all'esame critico delle disposizioni del provvedimento una pesante contestazione dell'attuale limitatezza del finanziamento statale delle università. Questa elencazione, ovviamente solo esemplificativa, evidenzia a sufficienza quanto sia stata e sia tuttora dura e intransigente la contrarietà dell'opposizione al provvedimento al nostro esame. Tale contrarietà, che a ben vedere riguarda solo alcuni contenuti del provvedimento, è stata ad arte strumentalmente estesa a tutto il provvedimento, per esacerbare ulteriormente l'attuale scontro politico, per contribuire alla "spallata" al Governo Berlusconi. Questo atteggiamento ha avuto purtroppo varie conseguenze negative. In primo luogo, esso è stato il riferimento e l'oggettivo sostegno di un movimento di fortissima protesta da parte di minoranze di studenti e ricercatori. Ne è derivata una sempre più grave lesione dell'immagine pubblica del provvedimento ed è stata resa impossibile la formazione di un ragionevole consenso, almeno nelle università. In questo stravolto contesto è esplosa nei giorni scorsi in varie città italiane, in particolare a Roma, una sconsiderata violenza di piazza. Di questo atteggiamento dell'opposizione ha sofferto anche l'esame parlamentare del provvedimento, che non ha potuto beneficiare appieno dell'importante apporto di una critica costruttiva. Verificheremo, signora Ministro, nei prossimi anni in che misura le numerose innovazioni del provvedimento conseguano effettivamente i loro obiettivi. non possono non seguire disposizioni di assestamento, di "*f**ine tuning*". A mio avviso andranno seguite con particolare attenzione la fondamentale innovazione dell'abilitazione scientifica nazionale e l'effettivo funzionamento dell'ANVUR, a cui il provvedimento affida un cospicuo carico di nuove incombenze, centrali per il buon funzionamento dei processi di valutazione della riforma. In conclusione, esprimo vivissimo apprezzamento per questo provvedimento, veramente di straordinaria importanza per la nostra università, certamente una delle tre o quattro grandi riforme di questa legislatura. Come hanno ben detto i colleghi del PdL che oggi mi hanno preceduto, vada avanti signora Ministro, senza paura. La strada imboccata è quella giusta!

giunti alle fasi conclusive di un *iter* lungo e complesso, com'era d'altronde inevitabile, data la complessità della materia. In questi lunghi mesi il disegno di legge è stato modificato e migliorato, arricchito di contenuti e snellito là dove era importante farlo. Sono stati infatti approvati numerosi emendamenti al Senato e alla Camera, anche dell'opposizione: a riprova di quanto il Governo ha sempre ribadito, cioè che siamo aperti ad ogni contributo migliorativo, purché nel solco dell'impianto riformista del provvedimento. Desidero in questa sede ringraziare tutti coloro che hanno dato un contributo di particolare importanza: il presidente Possa, il relatore, senatore Valditara, e tutti i componenti della 7a PdL),* nella quale, in prima lettura, abbiamo assistito ad un dibattito alto e appassionato, che ha contribuito in modo decisivo al miglioramento del testo. Oggi dobbiamo fare uno sforzo per completare il percorso del disegno di legge, per consentire al Paese e al suo sistema universitario di disporre di regole certe. Ricordo a tutti, dentro e fuori quest'Aula, che il sistema vive da tempo in un vuoto e in una incertezza normativa paralizzanti. Continuare a rimandare le decisioni significa solo lasciare persistere questo vuoto. È inevitabile che la dialettica parlamentare metta in evidenza le differenze anziché in punti di contatto, ma sappiamo che rispetto a tre mesi fa la situazione è diversa e migliore: i finanziamenti per il 2011 sono stati garantiti e sono adeguati. È giusto che, tolta questa ipoteca, oggi diamo il nostro assenso ad una riforma ordinamentale finalizzata a modernizzare i nostri atenei e a garantire che quei finanziamenti siano spesi al meglio. Sappiamo tutti altrettanto bene che la riforma del nostro sistema universitario è indispensabile e indifferibile. La documentazione sui suoi difetti strutturali è ampia e riflette posizioni politiche anche molto diverse tra loro. Non sono certo le diagnosi impietose a mancare: anzi, credo che troppo spesso le polemiche su alcune patologie pur gravi abbiano finito per oscurare i molti punti di forza dei nostri atenei e di coloro i quali in essi svolgono ricerca e didattica con passione e senso del dovere, tenendo alto il nome dell'Italia nel mondo della scienza e della cultura. Però, non possiamo neppure far finta, all'improvviso, che questa diagnosi, severa ed ampiamente condivisa, non esista, che tutto vada, in fondo, abbastanza bene, che non ci sia bisogno di un convinto sforzo riformista per migliorare. Solo perché una riforma è quasi arrivata in porto, anche se non sembrava, né facile, né forse neppure possibile, non possiamo tutto ad un tratto dire che è meglio lasciar perdere, che è meglio tenerci i problemi tanto lamentati,

vi parla, ma per le nostre università e per tutti coloro che da anni nutrono la speranza di un cambiamento; per gli studenti, i docenti, le famiglie; per quella grande maggioranza del Paese che non è andata in piazza, ma che merita di essere ascoltata. Il disegno di legge prospetta soluzioni di buonsenso a molti dei problemi che si sono accumulati negli anni. Non impone avventurose fughe in avanti né escogita utopie improbabili. Non è, non vuole essere, né reazionario né rivoluzionario. Auspico che prima di esprimere un giudizio tutti vogliano leggere attentamente il disegno di legge, senza pregiudizi, e giudicarlo per quello che è, e non invece come una pedina per uno scontro politico, pur legittimo, ma che non ha niente a che fare con i contenuti del disegno di legge Molti degli slogan che si leggono in questi giorni raccontano, lo dico senza spirito polemico, un disegno di legge che non esiste *(Applausi dal Gruppo di legge che regalerebbe l'università ai privati solo perché chiede che in consiglio di amministrazione siedano tre membri esterni, magari anche tutti professori di altri atenei, ma portatori di punti di vista meno direttamente coinvolti nelle vicende interne. Si parla di un disegno di legge che concentrerebbe tutto il potere nelle mani di pochi, anche se chiudiamo la strada a nuovi rettori a vita, limitando a sei soli anni, non prorogabili e non rinnovabili, il loro mandato, rendendo possibile la sfiducia e impedendo loro di continuare nella

si introduce finalmente una distinzione netta tra reclutamento e promozione, proprio perché sia più agevole la crescita professionale di chi se lo merita e si propone per la prima volta una seria programmazione pluriennale per i posti di professore. Che, infine, limiterebbe il diritto allo studio, proprio mentre il Governo non solo è riuscito a rifinanziare le borse di studio, ma ha anche fermamente respinto qualunque ipotesi di aumento, anche minimo, delle tasse universitarie, aumento che invece è stato Voglio fare chiarezza anche su un altro punto che ha suscitato ampie e, a mio parere, del tutto ingiustificate polemiche: quello relativo al finanziamento delle università telematiche. la pietra dello scandalo, è stato introdotto proprio al Senato senza suscitare alcuna critica. L'articolo si limita infatti a prevedere che una quota dei fondi statali alle università libere sia erogata non, come avvenuto finora, su base prevalentemente storica, ma sulla base di parametri di qualità uguali a quelli in uso già nel 2009 per il riparto della quota premiale del fondo di finanziamento (il famoso 7 La norma non aumenta e non diminuisce fondi per le non statali: prescrive solo che anche per esse debbano valere i criteri di valutazione della didattica e della ricerca previsti per le statali. Si tratta palesemente di una norma a favore del merito, che va incontro ad una richiesta da tempo avanzata proprio dalle università non statali. Le norme in vigore da anni prevedono già che a quei fondi possano accedere anche le università telematiche che abbiano superato due verifiche da parte del CNVSU, la prima dopo tre anni, la seconda dopo altri due. Aver stabilito criteri di qualità sulla base dei quali quei fondi saranno d'ora in poi distribuiti, non solo non rappresenta alcun favore fatto alle telematiche, ma anzi rende più difficile il finanziamento soprattutto per questo tipo di istituzioni, che sono anche le più giovani. Il nuovo regolamento sulle università telematiche, che intendo varare quanto prima, dimostrerà che il Governo intende agire per rafforzare la qualità di una parte importante del sistema universitario, senza sconti ma anche senza criminalizzarlo a priori. In queste ultime settimane il disegno di legge ha catalizzato una protesta giovanile diffusa, generazionale, che prescinde in molti casi dai contenuti specifici del provvedimento e segnala invece preoccupazioni e ansie che dobbiamo ascoltare con attenzione, purché siano espresse nel rispetto della legalità. Ma sappiamo tutti, onorevoli senatori, che gli studenti e i docenti hanno sempre protestato e protestano in modo civile. Le scene di guerriglia cui abbiamo purtroppo assistito non sono certo opera loro, ma di piccoli gruppi organizzati e violenti che non hanno certo a cuore le sorti della nostra università. Rispetto profondamente la legittima protesta dei giovani, ma non posso fare a meno di notare alcune strane analogie. anni fa, nel dicembre del 1989, nasceva il movimento della "Pantera", una protesta che per alcuni mesi paralizzò gli atenei italiani. Gli studenti temevano, allora come oggi, la privatizzazione dell'università, la morte dell'università pubblica, la fine della ricerca libera, soprattutto in campo umanistico; e qual era l'obiettivo di quella rivolta? Era la cosiddetta legge Ruberti sull'autonomia universitaria: quella legge la cui lungimiranza

Purtroppo, in alcuni momenti del passato recente questo disegno di legge è stato anche utilizzato come strumento di pura lotta politica. Oggi è nell'interesse del Parlamento e del Paese smorzare i toni, scendere dai tetti, abbandonare le polemiche, discutere meriti e limiti del provvedimento *(Applausi del senatore* *Possa)*. Il disegno di legge, ne sono profondamente convinta, segna un passo in avanti concreto, e mi sembra che, soprattutto negli ultimi tempi, quando sembrava in forse il suo destino, si sia iniziato a riconoscerne un po' più i pregi. Sono altrettanto convinta che anche le polemiche di queste ultime settimane si attenueranno una volta che apparirà chiaro a tutti in modo concreto che la nuova legge non stravolge il sistema universitario, che le nuove norme possono essere applicate subito, che si introducono miglioramenti importanti in molti settori della vita universitaria. Molte delle norme del disegno di legge prevedono già di poter essere superate, una volta raggiunti i risultati che ci attendiamo. Abbiamo avuto nei due anni scorsi la prova che, grazie a regole chiare e ad incentivi ben definiti, le università possono e vogliono cambiare. In due anni, grazie alle misure introdotte con la legge n. 1 del 2009 e ad una nuova consapevolezza delle proprie responsabilità, si è riequilibrato il rapporto tra ordinari, associati e ricercatori, superando quel modello a piramide rovesciata che costituiva un ostacolo enorme per le prospettive di carriera dei giovani accademici o aspiranti tali. Una fetta consistente del fondo di finanziamento ordinario è stato distribuita su base premiale, mettendo al centro della valutazione la qualità della ricerca. Sono già evidenti gli sforzi di moltissimi atenei per rafforzarsi in questa direzione e i miglioramenti che ne stanno conseguendo. Cambiare e migliorare, onorevoli senatori, è doveroso ma è anche concretamente possibile se si fissano obiettivi ragionevoli e traguardi sensati. Lasciatemi ricordare i principali punti di forza di questo provvedimento. Prima di tutto, l'accento posto sulla valutazione. Proprio grazie allo sviluppo di una pratica costante di valutazione ad ogni livello, dalla quale ci aspettiamo comportamenti orientati al merito, potremo un giorno, spero non lontano, superare quegli elementi di rigidità prescrittiva che il disegno di legge oggi necessariamente contiene. il sistema di ripartizione dei fondi pubblici basato sui costi standard e non sulla spesa storica (vera chiave di volta per superare sperequazioni storiche tra atenei); meccanismi di reclutamento, che si potranno spiegare al resto del mondo senza arrossire e che saranno finalmente in grado di attrarre studiosi anche dall'estero (oltre che, come spero, di trattenere i migliori cervelli nel nostro Paese). una *governance* meno pletorica e più responsabile, con una distinzione di compiti chiara tra il senato accademico e il consiglio d'amministrazione. Tutto questo inevitabilmente è troppo per alcuni e troppo poco per altri. Per me queste critiche di segno opposto sono la prova che ci siamo mossi con senso di responsabilità e rispetto, rifuggendo da pretese ideologiche ma anche rifiutando la facile strada dell'inerzia e della conservazione, cui pure ci esortavano in modo più o meno esplicito settori importanti della accademia che conta, poco interessati a cambiare abitudini consolidate. Come autorevolmente dichiarato stamattina dal professor Mario Monti, non solo il disegno di legge sull'università è un passo importante verso un sistema universitario più moderno e più funzionale, ma è una riforma che riduce la presa del sistema corporativo sull'università. Secondo Monti c'è bisogno di togliere un po' di potere a chi produce i servizi per darne di più a chi li deve ricevere: gli utenti e i consumatori. Per questa ragione, ha sottolineato Monti, la riforma va incontro agli interessi degli studenti. È una osservazione di una persona autorevole ed esperta di università che, credo, sia degna di nota. Altre soluzioni erano e restano possibili, è ovvio, ma molte delle soluzioni avanzate dal disegno di legge sono state ampiamente condivise nel tempo anche da una buona parte dell'opposizione. Penso all'abilitazione nazionale seguita da selezioni locali, le uniche che possono rendere un ateneo pienamente responsabile delle proprie scelte; penso al *tenure track*, che è la nuova disciplina su avanzamenti di carriera fondati sul merito. Penso alla centralità della valutazione. Le nuove regole sulla gestione della ricerca universitaria sono un esempio concreto di quanto fruttuosa possa essere la collaborazione tra maggioranza e opposizione quando si mette mano a problemi concreti con spirito costruttivo. All'emendamento proposto in quest'Aula dal senatore Marino sulla *peer review* si è aggiunto alla Camera quello della presidente Aprea che istituisce il comitato dei garanti per la ricerca. Questi due emendamenti sono complementari e si rafforzano a vicenda; spiace solo che questo metodo di lavoro non sia stato esteso ad altri aspetti della riforma. Al di là dei diversi ruoli che oggi siamo chiamati a svolgere, non possiamo ignorare questa base condivisa. Soprattutto, abbiamo il dovere di spiegare e far comprendere, di aiutare il sistema universitario a trovare serenità e normalità dopo le tensioni di queste ultime settimane. Nei prossimi mesi e anni metteremo alla prova questa legge e ne valuteremo con realismo pregi e difetti, rimanendo, come sempre, aperti all'ascolto, alla proposta e al confronto. Lo miglioreremo dove necessario e lo rafforzeremo, se ce ne sarà bisogno, ma non diciamo neppure per scherzo che è meglio ritirare il disegno di legge e riaprire una discussione infinita, sostenendo magari che l'*iter* del provvedimento è stato eccessivamente frettoloso. Ricordiamoci alcuni fatti concreti: le linea guida del Governo sull'università risalgono all'autunno del 2008; una stesura quasi definitiva del disegno di legge era stata illustrata a tutti i rettori nel marzo 2009, per essere poi presentata al Senato nell'ottobre dello stesso anno. La 7a Commissione permanente del Senato ha condotto decine di audizioni prima di esaminare oltre 800 emendamenti, discutendoli uno per uno senza alcuna limitazione dei tempi. Altri 500 emendamenti sono stati discussi e votati in Aula al Senato e poi ancora mille tra Commissione e Aula alla Camera. Chiamare frettoloso questo lavoro certosino significa disconoscere l'enorme impegno parlamentare che lo ha reso possibile. So bene che la richiesta più forte che ci viene soprattutto dai giovani studiosi è quella di rimettere in moto un meccanismo inceppato e di evitare nuovi ritardi. Voglio tranquillizzarli: con la nuova normativa, gli assegni di ricerca potranno essere banditi all'indomani dell'entrata in vigore della legge senza alcun intervento regolamentare o normativo. Lo stesso vale per i posti da ricercatore, per i quali il disegno di legge richiede solo un semplice regolamento di ateneo. Ribadisco solennemente in questa Aula l'impegno a far uscire i provvedimenti applicativi di cui è responsabile il Ministero nel più breve tempo possibile, partendo da quelli indispensabili per mettere in moto le procedure di abilitazione e di chiamata. Sui provvedimenti di attuazione del disegno di legge si gioca, come tutti sappiamo, una partita molto importante. Mi auguro con convinzione che su questi provvedimenti, anche al di là dei meccanismi formali, si apra un confronto costruttivo con tutte le forze che hanno a cuore il futuro della nostra università. Sarebbe del tutto incomprensibile estendere anche a questa fase del lavoro un clima di contrasto, che è invece nell'interesse di tutti (soprattutto degli studenti, dei docenti e degli atenei stessi) archiviare una volta approvata la legge. Rinnovo quindi il mio caloroso invito anche all'opposizione perché non faccia mancare il suo contributo. De Gasperi ebbe ad affermare: «Chi governa deve guardare alle prossime generazioni». Questa riforma è, e resta, per i ragazzi di oggi e di domani. Bisogna avere il coraggio di cambiare, e sono certa che questa Assemblea vorrà dimostrarlo: vorrà dimostrare di avere fino in fondo il coraggio di puntare su una università

un *iter* brevissimo durato circa 48 ore. Il presidente Possa però non ha riferito alcuni accadimenti destinati, a nostro modo di vedere, ad incidere sul prosieguo dei lavori,

Il presidente Possa rispose affermando testualmente: «Non occorre aspettare i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, fermo restando che essi sono resi per l'Aula, poiché il provvedimento è calendarizzato in Assemblea» La tesi del presidente Possa è cioè che nel momento in cui la Conferenza dei Capigruppo calendarizza un provvedimento in Aula, la Commissione di merito può fare a meno dei pareri della 5a e della 1a Commissione: un'affermazione questa palesemente contraria al nostro Regolamento e certamente alla prassi, mai da nessuno messa in discussione, che si è determinata. Nella seduta pomeridiana, signor Presidente, sempre il nostro Capogruppo, dopo aver constatato che la 5a Commissione non era stata neanche convocata per potere esprimere i pareri stessi, ripropose il tema e propose una questione sospensiva del Regolamento, rigettò questa questione non ponendola neanche ai voti, sostenendo che la stessa questione sospensiva non era

e noi tutti sappiamo, che in questo caso non è affatto applicabile l'articolo 93 del nostro Regolamento, che riguarda appunto i lavori ma è applicabile un'altra norma specifica, contenuta nel nostro Regolamento, l'articolo 43, comma 3, che tratta la questione delle sospensive in Commissione e non pone alcun limite temporale alla proposizione di quelle questioni in Commissione. Tanto più che, come nel caso che ci occupa, che la questione posta dal senatore Rusconi era sopravvenuta, cioè si stava verificando in quelle ore il fatto che la Commissione di merito aveva iniziato a votare gli emendamenti in Commissione senza il parere della 1a e, soprattutto, senza il parere della 5a Commissione. Nella seduta pomeridiana, iniziata se non ricordo male, attorno alle 15, prima delle ore 17, sempre il Presidente Possa, dopo aver constatato ore erano stati votati 35 emendamenti, come egli stesso ha riferito questa mattina, ha chiesto ai Gruppi presenti il da farsi, e le cose sono andate come lui ha riferito e come ha confermato questa mattina il senatore Rusconi. Cioè, ci fu una disponibilità da parte del nostro Gruppo (e non solo del nostro) a rinunciare a una parte consistente - anzi, alla gran parte - degli emendamenti, ove vi fosse stato un atteggiamento di apertura da parte della maggioranza. Dopo aver verificato che questo atteggiamento di apertura, per espressa dichiarazione dei Gruppi di maggioranza, non c'era, si chiese di poter procedere all'esame degli emendamenti. Sennonché il presidente Possa, apprezzate le circostanze, alle ore 17, dopo aver appena iniziato l'esame della Commissione...

il diritto di sciogliere la seduta della Commissione giovedì pomeriggio, dopo 48 ore circa dall'inizio dell'esame di un provvedimento così complesso, difficile, discusso e contrastato,

non lo possiamo accettare perché si tratta di un modo di condurre i lavori che si pone in palese contrasto con l'articolo 72 della Costituzione,

sappiamo tutti che l'aspetto finanziario era - ed è - uno dei più controversi per questo provvedimento. Per queste ragioni signor Presidente, credo che sarebbe saggio, saggio, serio e lungimirante che la maggioranza accedesse alla richiesta che noi formuliamo di non passare all'esame degli articoli, di rimandare il testo in Commissione, di far lavorare la Commissione e di calendarizzare il provvedimento in una data certa. Non c'è alcuna istanza da parte nostra, così come non c'è mai stata, di un rinvio *sine die*.

faccia le proposte. Noi le abbiamo fatte e le stiamo facendo: vogliamo lavorare, esaminare e coltivare questo confronto. Da parte vostra non c'è stato, fino a questo momento, alcun segno di voler concretamente attuare quello che lei, signora Ministro, a nome del Governo, ci ha detto. Per queste ragioni, nel caso voi non riteniate di accogliere questa nostra ragionevole proposta, che aiuterebbe anche ad allentare la tensione che vi è nel Paese rispetto a questo

Questo è ciò che è avvenuto. Molto semplicemente, noi siamo contrari alla proposta del senatore Legnini. [LI Signor Presidente, onorevoli colleghi,

l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto che il Senato avesse commesso 55 errori, tant'è vero che ha apportato 55 modifiche al testo licenziato da quest'Assemblea.

che un disegno di legge di questa importanza, che l'altra Camera corregge in 55 punti, non possa essere approfondito attraverso l'esame in Commissione, per verificare se quelle 55 modifiche al nostro lavoro abbiano un loro fondamento? Lo

il valore di questa Camera Alta della Repubblica! Non accettiamo che ci vengano imposti compitini senza poter più discutere neanche una virgola. Ritengo quindi che la proposta del collega Legnini abbia un fondamento, non solo nel merito merito e nel metodo, ma perché rivendica a quest'Aula le sue alte prerogative, nel senso che siamo in grado di correggere, come abbiamo fatto in tante altre occasioni, ciò che viene dall'altro ramo del Parlamento.

Secondo dato. Stamattina ho ringraziato il Presidente per la sua correttezza, perché quando i Gruppi del PD e dell'Italia dei Valori hanno chiesto di approvare tre emendamenti di merito non hanno ritenuto gli altri ininfluenti, hanno chiesto al Governo la disponibilità a entrare nel merito del diritto allo studio, nonché una disponibilità rispetto al dato dei ricercatori. Di fatto, però, la risposta è stata che il disegno di legge è immodificabile. Rispetto a questo, non so da quale parte stia l'ostruzionismo o la disponibilità a dialogare.

della collega Garavaglia di cominciare i lavori alle ore 15,30 per poter permettere ad alcuni colleghi di assistere alla messa

I colleghi dell'opposizione hanno posto una questione che dal punto di vista politico e della loro prospettiva, non avendo votato il calendario, è corretta. Peraltro, corrisponde al vero che il testo

era giusto che fossero oggetto di esame e di approfondimento sia in Commissione che in Aula. Per quanto riguarda il nostro Gruppo parlamentare, poiché abbiamo votato il calendario che prevedeva l'impegno

comuni con altri Gruppi parlamentari di opposizione, che si trasformeranno in un ordine del giorno, circa il cronoprogramma di attuazione della riforma. Queste sono le ragioni che, pur dando atto ai colleghi del PD e dell'Italia dei Valori di aver posto una questione corretta, ci portano a non poter aderire alla loro richiesta e quindi a non votare

Presidente, a noi piace sempre guardare in faccia la realtà e dire come stanno le cose.

Io vorrei leggere alcune righe di un testo, che poi vi renderò noto, che così recita: «Dobbiamo avere il coraggio di affermare che i fondi devono essere spesi in un altro modo. Questa università, così com'è, non ci piace e non funziona. È una università in cui si va avanti ancora con logiche di tipo baronale, di mantenimento di piccoli spazi, in cui molti insegnanti non fanno lezioni e non sono a disposizione degli studenti, non dialogano con loro e non fanno ricerca». Apparentemente, questo potrebbe essere un testo attribuibile al ministro Gelmini, visto che ella incardina su questi difetti la riforma dell'università. Ahimé, questo non è un testo

due spiegazioni circa le modalità di gestione dei lavori della Commissione in questi giorni.

5a. Naturalmente, io chiedo sempre agli uffici che mi affiancano se il procedere

emendative. Nel momento in cui abbiamo ricevuto un rifiuto da parte del Governo, abbiamo detto che non intendevamo ritirare i nostri emendamenti. A questo punto, la maggioranza ha concluso che, visti i tempi impiegati (circa quattro ore in Commissione),

Grazie, D'altra parte, questo significherebbe che della metà del lavoro che fanno la Commissione bilancio e la Commissione affari si potrebbe fare a meno. È vero questo? Si pronunci la Giunta per il Regolamento. Il secondo punto, sempre sulla Giunta per il Regolamento, ci sarebbero numerosissimi precedenti circa l'applicabilità dell'articolo 93 ai lavori di Commissione. Io non so quali siano questi precedenti, vorrei conoscerli, ma temo che non ci siano, per la ragione che, come ho già detto nel mio precedente intervento, vi è una norma espressa sulle questioni sospensive in Commissione (l'articolo 93 riguarda i lavori questa norma, l'articolo 43, terzo comma, dice: «In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive». La norma aggiunge: «Ove siano avanzate» - in tal modo affermando che possono essere avanzate

perché è evidente che, ove proposte, queste questioni non determinerebbero lo stesso effetto previsto dall'articolo 93 per i lavori d'Aula, cioè quello di arrestare l'esame del provvedimento, ma una questione una questione sospensiva in Commissione produrrebbe, ove approvata, l'obbligo di riferire all'Assemblea per le determinazioni del caso. È quindi evidente che quel richiamo all'articolo 93, fatto sulla base di presunti numerosi precedenti, è assolutamente

accettata dalla maggioranza, anche con il voto di poco fa, significherebbe - lo ripeto -stravolgere i lavori del Senato di qui in avanti, e questo noi non lo possiamo accettare. finestra"). È del tutto evidente, senatore Legnini, che per assoluta correttezza di ruoli riferirò al presidente Schifani questa sua posizione. Devo dire anche, con altrettanta chiarezza, che raccomanderò al presidente Schifani di fare questa valutazione nella Giunta del Regolamento, perché non c'entra niente in questo caso la conduzione punti ambigui o comunque non chiariti nell'interpretazione del Regolamento, è bene che siano chiariti. Quando tra l'altro nella Conferenza dei Capigruppo si prende la decisione di porre all'ordine del giorno dell'Aula un provvedimento, a volte serve anche per dare una scadenza al lavoro delle Commissioni,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere, nei casi delle università il cui

mi sembra strano che il Governo, una volta cambiato il Ministro, che adesso fa parte di un partito che non sostiene più questa maggioranza, si dimentichi tutto quello che ha fatto fino ad oggi. Stiamo parlando di due

per dottorandi, ricercatori o professori non abbiano carattere discriminatorio; a garantire comunque - questa sarebbe una questione più generale - un adeguato sistema permanente e pubblico di monitoraggio e di valutazione dello stato di salute della lingua nazionale. Questo, anche perché una delle poche fonti di introito per le nostre ambasciate o istituti di cultura nel mondo è per l'appunto l'insegnamento della lingua italiana, che sta conoscendo una nuova primavera, all'estero e non in Italia. Non si riesce dunque a comprendere il motivo per cui sia stato espresso parere negativo su questo ordine del giorno, che si inseriva in un filone di tutela e promozione della nostra lingua che il Governo, fino alla settimana scorsa, aveva portato avanti. Qualora non dovesse esserci la

signore e signori del Senato, il collega Perduca pretende con questo ordine del giorno, che chiede sia votato, visto che c'è un parere negativo del Governo, che che i laureandi in lingue straniere, vuoi inglese, vuoi francese, tedesco o cinese, abbiano il diritto di redigere la loro tesi di laurea

ed a garantire ad ogni cittadino residente in Italia» - a parte che non si capisce perché "cittadino" - «il diritto di seguire gli insegnamenti, sostenere gli esami, partecipare ai concorsi, redigere la tesi di laurea e/o di dottorato o insegnare, in lingua italiana». Una bella insalata russa. Grazie,

Grazie, signor Presidente. Volevo dire che gli uffici non hanno sufficientemente studiato quanto quest'ordine del giorno possa influire, per esempio, sulle competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. Per quanto riguarda l'articolo 29, comma 22, in relazione all'assenza di una clausola di salvaguardia, valutato che: per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo 22, i parametri adottati nella quantificazione conducono ad una sovrastima significativa dell'onere, tanto da ritenere che la clausola di salvaguardia anche qualora fosse stata prevista non sarebbe presumibilmente stata operante nella sostanza; e che il comma 7 del medesimo articolo 22 prevede un meccanismo di modulazione degli oneri suindicati, posto che consente al soggetto che conferisce l'assegno di determinare l'importo dello stesso sulla base di un importo minimo stabilito con decreto, esprime, tuttavia, parere di semplice contrarietà. Osserva, inoltre, la necessità di rendere compatibile e trasparente il sistema contabile delle università, anche attraverso appositi schemi di raccordo tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale secondo quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009. Occorre inoltre che, in relazione ai contratti di apprendistato, l'indizione delle procedure avvenga solo nel limite delle risorse disponibili degli atenei». degli atenei». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 2.23, 2.25, 2.120, 2.305, 2.308, 4.18, 4.302, 4.307, 5.30, 5.31, 5.32, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.315, 6.16, 6.304, 6.306, 6.315, 19.7, 19.306, 19.308, 19.12, 21.304, 21.321, 21.324, 21.325, 22.317, 22.318, 22.321, 23.27, 23.346, 24.16, 24.300, 24.303, 29.324, 29.325, 29.327, 29.328, 29.329, 29.28, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 5.311, 5.316, 5.317, 22.309, 23.343, 24.304 e 24.305. Sugli emendamenti 2.309 e 3.0.1, il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia inserita una clausola d'invarianza degli oneri». Onorevoli colleghi, poiché, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, il Senato discute e delibera solo sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, dichiaro inammissibili gli emendamenti 1.302, 2.308, 2.306, 2.309, 2.312, 3.0.1, 4.26, 4.27, 4.330, 4.37, 4.334, 5.4, 5.8, 5.9, 5.46, 6.304, 6.305, 6.306, 6.318, 11.300, 23.346, 24.303, 24.304, 24.305, 25.300, 25.301, 25.302, 25.303,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stata qui evocata poco fa la necessità di migliorare l'insegnamento della lingua italiana. Forse, questo invito è meno teorico e peregrino di quanto si possa pensare: negli emendamenti che la Camera ci ha presentato l'elemento fondamentale che ritorna sempre, e il tema consueto che si ripete nella sequenza di tutti gli articoli, è una straordinaria mancanza di chiarezza degli enunciati, che ci pone certe volte nella difficoltà di capire le intenzioni, e una certa tendenza alla farraginosità e alla complicazione. Gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 fanno, in realtà, riferimento a difficoltà generate dalla

a ritornare alla formulazione originaria, anche perché il sottofondo che emerge dall'analisi del testo fa pensare che, con queste modifiche

come è già stato osservato nella discussione in Commissione - la Repubblica è composta da Comuni, Province e Regioni e, nel momento in cui si scrive «al sistema universitario della Repubblica» si crea, in realtà, una confusione non necessaria. Allora, la nostra proposta nell'emendamento 1.7 è di sostituire le parole: «al sistema universitario della Repubblica» con le seguenti: «al pubblico sistema universitario». Ciò cancellerebbe le possibili confusioni generate dall'uso del termine "universitario della Repubblica" e inserisce volontariamente il il peso dell'aggettivo "pubblico" perché noi abbiamo profondamente a cuore che il sistema universitario si caratterizzi sempre e costantemente per il valore dell'azione pubblica, e perché ci teniamo che la scuola e l'università siano un patrimonio pubblico e non privato. privato. Nella formulazione precedente, invece, nulla esclude che nel sistema universitario della Repubblica si possano considerare anche le università private.

resi necessari da una confusione del testo che francamente rende preferibile il ritorno alla formulazione precedente. Sottolineo,

Quindi, siamo di fronte alla necessità di una correzione obiettiva. Il punto più importante degli interventi emendativi all'articolo 1, onorevoli colleghi, su cui attraggo la vostra attenzione, è che

in Aula - che «Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse ed il Ministero, al fine di favorire la competitività delle università svantaggiate,»

Grazie a... non so che cosa, si potrebbe dire! Dove sta il grande significato di questa frase?

si possano fare delle deroghe. Si dice testualmente: «ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica,

prevede l'introduzione di un termine entro cui il Ministero deve comunicare alle università qual è la quota del fondo che viene loro assegnata. L'obiettivo è di dare certezza alle università di poter fare i bilanci e - comunque - di poterli predisporre entro l'esercizio finanziario. Ci rendiamo conto che la quantità di risorse legge di stabilità e, per quanto tale legge possa avere, a seguito della riforma, tempi molto più brevi della vecchia legge finanziaria, l'emendamento non prevede che debba essere quantificata entro il 31 ottobre l'entità

che le procedure e le valutazioni degli atenei vengano fatte in termini oggettivi, e non in ragione delle quantità di risorse che ogni anno la legge di stabilità trasferisce al Ministero. Ripeto: se il Governo ritiene

policentrica indica qualcosa che potrebbe funzionare come un centro polifunzionale policentrico, un'attività culturale,

il valore del sistema pubblico. L'università pubblica, la scuola pubblica hanno un carattere centrale nella Repubblica italiana.

dei meno abbienti e deve rimuovere gli ostacoli che si frappongono al compimento della personalità umana.

cui facciamo riferimento è e deve essere pubblica e l'università privata, se esiste, deve camminare con le proprie gambe, i propri finanziamenti, le proprie energie, senza concessioni al raggiungimento di facili profitti che, tra l'altro, introducono nuove diseguaglianze. Si tratta quindi di un emendamento profondamente incardinato sull'idea dell'eguaglianza.

le università dello Stato, quindi le università pubbliche, debbano avere comunque un'assoluta considerazione e una priorità, sia riguardo al sistema di finanziamenti che a quello di una riforma ordinamentale che le coinvolge pesantemente. Credo che sia ancor più appropriato dire «università dello Stato» ma, comunque, voteremo a favore di entrambi gli emendamenti, anche perché corrispondono a una proposta che, per primi, abbiamo presentato in quest'Aula e che, purtroppo, allora non ha visto neanche il conforto

un vero e proprio atto di forza, incurante del clima di particolare tensione che la riforma sta generando, clima causato dall'arroganza del Ministro e della sua coalizione, che non hanno inteso ascoltare né gli studenti, né i ricercatori, né tutti i precari, che vengono sacrificati da una legge sbagliata e iniqua. Massacrare la ricerca e l'università pubblica è fuori da ogni logica e va contro l'interesse del Paese. Non si può pensare che l'asse Tremonti-Gelmini pretenda di riformare l'università senza adeguati investimenti che, esaltando il merito, diano la possibilità agli studenti meritevoli, e anche a chi non ha le risorse, di proseguire gli studi. Dopo aver provato a camuffare i tagli al comparto cultura, alle fondazioni liriche, alla scuola pubblica, al sostegno al patrimonio culturale, ora questa riforma celebra il *de profundis* anche dell'università. Considerare la ricerca un inutile orpello dimostra la volontà di tagliare il futuro dei giovani e, quindi, del Paese. Oggi, signori del Governo, blindate questo provvedimento come state cercando di blindare i Palazzi del potere da una contestazione legittima, che i gesti di un manipolo di violenti

di concreto, non dice molto, ma contiene i principi ispiratori della riforma. Signor Presidente, se noi dai principi ispiratori eliminiamo

PdL).* L'ostruzionismo parlamentare lo fate voi, perché nel momento in cui il Parlamento non è nelle condizioni di dialogare, discutere e modificare neppure una virgola,

trattazione farò notare, ci rendiamo conto che qui c'è una volontà esplicita di promuovere un federalismo culturale, cioè sostanzialmente di regionalizzare le università, dicendo che i livelli essenziali delle prestazioni li garantisce, sì e no, lo Stato: poi, se i privati e le Regioni lo vogliono,

significa avere come principio ispiratore un'idea di università che tradisce profondamente l'articolo 3 della Costituzione. Chiedo per questa ragione, signor Presidente, il voto elettronico, perché ogni collega deve prendersi la responsabilità di spiegare poi sul territorio come ha votato su questo emendamento.

di arrivare ad una rapida approvazione è dovuta anche ad una considerazione politica. Sono necessari decreti attuativi, e penso che le le università non possano ancora aspettare, come succederebbe se il testo venisse rinviato alla Camera. Condivido l'aspetto politico delle motivazioni esposte dal senatore Procacci,

La differenza fra chi è professore e parla con gli studenti indisciplinati e gli avvocati che parlano invece in aule silenziose è che io riesco a parlare lo stesso,

che chiunque abbia esperienza amministrativa sa che rende difficile l'applicazione o addirittura crea l'alibi per non fare quanto la norma detta. Si fa riferimento alla determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane. Ad un certo punto si parla anche dei posti vacanti e, al «Il posto che si rende in tal modo vacante può essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni». Ma come "può"? Se ci sono disposizioni vigenti in materia di assunzione, non Abbiamo sentito, tutto il pomeriggio, citare la necessità della chiarezza e della trasparenza della normativa affinché questa sia attuabile.

la competenza del senato accademico e la composizione del consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia la durata del mandato del rettore, con l'emendamento 2.26 si ripristina

alla Camera la possibilità di due mandati di quattro anni non superiori agli otto anni, ed essendoci quindi un unico mandato di sei anni, dire che occorrono due terzi per la sfiducia significa rendere tutto più rigido. Pertanto,